Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, la situazione nelle carceri italiane è grave e insostenibile, sia dal punto di vista delle condizioni sanitarie e trattamentali, per quasi la totalità. Il tempo trascorre nell'ozio, in condizioni di promiscuità e igienico-sanitarie spesso oltre il limite di ogni decenza, senza attività di rieducazione, di lavoro, di altra azione formativa. Ricordo che il numero di soggetti dediti alle varie forme di lavoro non supera il 15 per cento degli appartenenti alla popolazione carceraria. L'emergenza che caratterizza questa nostra situazione deriva da un ritardo storico nell'adeguamento delle strutture in termini di quantità di posti disponibili, ma anche, e non ultimo, di qualità degli ambienti e di inadeguatezza degli stessi per il raggiungimento delle finalità rieducative. Una questione di grande rilievo è rappresentata dalla convinzione, culturalmente radicata nell'opinione pubblica, in una parte degli operatori del diritto e anche nel legislatore del passato, che l'unica sanzione vera è quella detentiva che ad essa sola è affidata un'azione deterrente concreta da parte del nostro ordinamento penale. Un grandissimo ritardo nell'affrontare il problema con un'adeguata azione di depenalizzazione ha provocato certamente una situazione ormai di ingestibilità. L'alleggerimento dell'emergenza attraverso una vera azione di depenalizzazione avrebbe comportato una maggiore selezione e più efficacia nell'azione di deterrenza, che oggi si manifesta in maniera molto limitata, proprio perché c'è un atteggiamento di comprensione della situazione carceraria, per cui molti provvedimenti vengono assunti proprio tenendo conto di questa particolare situazione di insostenibilità. È necessario quindi affidare ad un'azione di tipo straordinario il ripristino di un minimo di legalità all'interno del nostro sistema carcerario rispetto, quanto meno, ai principi fondamentali dei diritti umani.

misure di un certo peso e dettate anche da una certa preoccupazione, proprio perché la situazione è diventata insostenibile.

Certo, competerà ai tribunali di sorveglianza il compito di rispondere tempestivamente e appieno ai dettami di questo nuovo provvedimento.

altrimenti la misura non avrebbe inciso in maniera significativa sul numero degli ospiti del nostro sistema carcerario. Non dobbiamo dimenticare, però, che nell'opinione pubblica c'è un certo allarme, che si presta anche a qualche strumentalizzazione da parte delle forze politiche che in questi anni, sull'argomento della sicurezza dei cittadini, hanno fatto e disfatto a loro piacimento, quando erano all'opposizione e quando erano al Governo. Quindi, ci aspettavamo non l'accoglimento dell'ordine del giorno sulle questioni sottese ai nostri emendamenti 1.208 e 1.216, ma una risposta puntuale, che invece non abbiamo avuto.

Non è vero, signor rappresentante del Governo, che la materia è adeguatamente trattata nella nostra normativa vigente, perché allora mi si deve spiegare per quale ragione

È evidente che c'è qualcosa che non funziona nell'attuale normativa. In particolare, la possibilità dell'utilizzo dei braccialetti elettronici soltanto a fronte della disponibilità del detenuto rappresenta un limite. Non c'è, da parte del magistrato che deve applicare la disposizione della detenzione domiciliare, la possibilità di esercitare una sorta di trattativa: o accetti il braccialetto o rimani in carcere.

notizie che abbiamo circa 50.000 carcerabili utilizzano il sistema del controllo con il braccialetto elettronico.

Con questa presenza avremmo potuto rassicurare l'opinione pubblica ed anche alleggerire il lavoro oneroso che in questo caso, invece, viene assegnato alle forze dell'ordine, i cui rappresentanti oltre a svolgere la necessaria azione di prevenzione e di repressione dei reati, devono far

Si sarebbe realizzato anche un grande risparmio. È evidente, infatti, che il mantenimento di una persona in carcere, rispetto al mantenimento di una persona presso presso la propria abitazione, riducendo al minimo il sistema di controllo fisico sostituito da quello elettronico, avrebbe certamente ridimensionato i costi relativi alla detenzione.

e introducendo anche quelle eccezioni che sono necessarie per salvaguardare comunque l'opinione pubblica e i cittadini da pericoli che potrebbero derivare da reimmissioni, non in libertà ma in detenzione meno controllata e rispetto a alcune fattispecie di comportamenti che sicuramente possono rappresentare un fattore di preoccupazione. Per queste ragioni, esprimiamo il nostro voto favorevole al provvedimento, con l'auspicio che il futuro possa essere di maggiore attenzione rispetto alle problematiche che abbiamo richiamato. Signora Presidente, signor Sottosegretario, «per me si va ne la città dolente, per me si va ne l'etterno dolore, per me si va tra la perduta gente»: questi sono famosi versi danteschi della Divina Commedia.

terribilmente; accompagnato da Virgilio, il poeta ovviamente entra nell'Inferno, città del dolore e della pena. Questi versi, letti da studente e da legislatore, cari

che differenza c'è quando, per carcerazione preventiva (il 43 per cento, 26.000 persone) o per espiazione di una di una pena per una sentenza passata in giudicato (41.000 persone), degli umani varcano la porta del carcere? Oggi come allora si va nella città dolente, si va nell'eterno dolore, si va tra la perduta gente; e oggi come allora

che causano patologie e alterazioni organico-funzionali in un numero di dieci-venti volte superiore alla media nazionale; una vera e propria pandemia carceraria, tra tubercolosi, micosi, epatite B e C, virus della mononucleosi, tifo e paratifo, parassitosi, malattie esotiche, esotiche, comprese autolesioni, ferite e traumi provocati da atti di violenza, con suicidi (60 nel 2012 un dato dieci volte superiore alla media nazionale), omicidi, senza contare le violenze sessuali. Sì, anche quelle; c'è qualche pm o giudice che lo fa proprio apposta nel favorire e permettere questo. Una volta che queste persone, pagato il debito ma non rieducate, ritornano a casa, diventano dei veri e propri untori di manzoniana memoria.

lì per essere rieducati, ma a soffrire, a essere torturati, senza che venga loro riconosciuta la forma più elementare di dignità e di speranza per loro stessi, per la loro famiglia e per il loro futuro reinserimento lavorativo e sociale.

Non è tortura, in queste condizioni, sapendo che 13.000 di quei 26.000 detenuti in attesa di giudizio saranno giudicati un po' di tempo dopo innocenti? Ma se un medico sbagliasse un'operazione, cosa gli fareste? Perché un giudice ne può sbagliare dieci, cento, mille e nessuno gli fa

che, per loro bramosia personale, portano in carcere, abbiamo detto, addirittura 13.000 persone innocenti. Gli esempi li conoscete: Di Pietro, Ingroia, De Magistris e altri. le sentenze Tortora, Pacciani, Andreotti (di Perugia o Palermo), di Craxi, di Forlani, di Del Turco, degli scienziati dell'Aquila, di

(è un termine sanscrito della religione induista, che è positivo, mentre qui è solamente sinonimo di cattivi maestri

se non il figlio calabrese di un operaio; a quei *guru* che portano alla ribellione i No TAV, con implicato anche il figlio di un giudice. Ebbene colleghi, i fatti e i numeri dicono che penitenziari italiani sono sono colmi, in barba a quanto previsto dalla nostra stessa legislazione, che rischia di non trovare piena e concreta applicazione dinanzi al fenomeno del sovraffollamento. Ciò ci espone a sanzioni da parte della Corte di Strasburgo, che in più occasioni ha già imposto allo Stato italiano il risarcimento dei danni morali in favore dei detenuti ai quali non erano assicurati gli *standard* minimi presso i penitenziari cui erano assegnati. Vi leggo anche i numeri della nostra Costituzione: articolo 13, comma articolo 32, comma uno. Poi ricordo l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché la legge sull'ordinamento penitenziario n. 354 del 1975. Perché così tante leggi disattese? Le previsioni che allargano la quota della popolazione carceraria che può essere destinata a lavori di pubblica utilità nei campi sociali della sanità e del volontariato costituiscono un passo avanti importante per quanto attiene al ruolo rieducativo e riabilitativo della pena. È per questo che noi, come Gruppo, diamo un giudizio positivo. Perché un po' è meglio che niente. Perché compito dello Stato è quello di garantire il pieno rispetto dei diritti di tutti i suoi cittadini, detenuti compresi. Se l'attuale condizione carceraria non consente il rispetto di tali diritti, allora è indispensabile provvedere con misure alternative, come la liberazione anticipata o la detenzione domiciliare, contenute nel provvedimento in esame. Se i diritti dei detenuti non sono garantiti è infatti lo stesso Stato a delinquere nel momento in cui non è in grado di assicurare il rispetto delle sue stesse leggi. Questo non è accettabile. L'articolo 608

E questo non perché lo dica io, ma alla luce delle richiamate sanzioni e raccomandazioni ricevute dall'Europa. Ricordo anche diversi appelli rivolti al Parlamento in questi anni dal Capo dello Stato, nonché da svariati esponenti dei diversi Governi che si sono succeduti nelle due scorse legislature. Certamente le misure contenute in questo decreto non saranno sufficienti. Certo, quello del Governo è un buon testo, che il Senato ha contribuito ulteriormente a migliorare, sia in Commissione che in Aula, anche grazie all'atteggiamento non preclusivo tenuto dall'Esecutivo, per il quale vorrei ringraziare il

il decreto sulle carceri varato dal Governo è, ad avviso della componente Sinistra Ecologia e Libertà del Gruppo Misto, un passo in avanti sulla via di un ritorno alla civiltà, dalla quale il nostro Paese negli ultimi anni si è di molto allontanato. Il solo motivo di rammarico, l'ho già detto ieri, è che questo passo sia stato mosso in seguito ad una direttiva europea stringente e non come una scelta autonoma e responsabile di una politica capace di rimediare ai propri errori. Riconosciamo al Governo di non essersi limitato a varare norme in uscita, tanto per fare un po' di spazio in più nelle patrie galere, ma di essere intervenuto anche in entrata, favorendo il ricorso alle misure alternative alla detenzione per i casi meno gravi e per i detenuti in attesa di giudizio, che rappresentano ‑ come sappiamo ‑ la netta maggioranza della popolazione carceraria. Consideriamo questo un passo avanti, sicuramente, ma non sufficiente. Per uscire infatti dalla dimensione di inciviltà nella quale versano le nostre carceri bisogna fare molto di più, anche alla luce del fatto che avremmo voluto vedere in quest'Aula non più coraggio, come qualche volta si dice, ma più senso di responsabilità, in particolare rispetto ad alcune questioni, come quelle relative ai tossicodipendenti, sulle quali si doveva e si poteva intervenire molto meglio. Occorre, secondo noi, cancellare le leggi criminogene che sono state adottate in questi anni, come quelle sull'immigrazione e sugli stupefacenti, e che sono state uno dei motivi del sovraffollamento:

Pensiamo insomma che si debba ribaltare l'idea di fondo che c'è stata nel corso di questi anni e che è stata portata avanti dai Governi di centrodestra innanzitutto, ma purtroppo troppe volte avallata anche dalle forze politiche del centrosinistra, colpevole dal nostro punto di vista di avere completamente rimosso quel poco di storicamente già assai debole cultura garantista, sacrificata con totale disinvoltura sulla base di qualche calcolo elettorale. La costruzione di un immaginario che faceva diventare l'ossessione securitaria la leva per contrastare le paure e le insicurezze sociali generate dalla crisi è diventato il potentissimo retroterra culturale con il quale abbiamo dovuto convivere e confrontarci. se abbiamo chiamato tutto questo «fabbrica della paura» è perché abbiamo avuto l'impressione che questo retroterrra, questo immaginario fosse utilizzato come una vera e propria arma di distrazione di massa, tesa a costruire un universo di valori e una scala di priorità la sicurezza, innanzitutto, o presunta tale - rispetto alla quale dovessero fare un passo indietro anche quei diritti individuali conquistati dopo anni di battaglie civili e sui diritti umani. Si pensi, Presidente, alla legislazione di questi anni. Nello stesso momento in cui si varavano le leggi *ad personam* e i vari lodi tesi ad assicurare le più totali garanzie ad esempio per il Presidente del Consiglio, si costruiva un poderoso assetto culturale capace di stravolgere finanche alcune garanzie contenute nella Costituzione repubblicana e si sventravano leggi, come la Gozzini, che avevano rappresentato una speranza di interrompere il perverso meccanismo delle porte girevoli, secondo il quale la possibilità per un detenuto uscito di galera di tornarci è altissima. E si passava in definitiva, con il consenso di tanta parte della popolazione, sedotta dalla retorica feroce della punizione, da uno Stato sociale ad uno Stato penale. È stata, a nostro avviso, una vera e propria doppia morale quella contro la quale ci siamo dovuti battere, spesso in solitudine, legata alla difficoltà di far vivere questi temi in un'opinione pubblica molto condizionata anche dalle posizioni politiche - come già ho avuto modo di dire - di una parte consistente della sinistra italiana. Si pensi ad una legge manifesto di questa ideologia, la ex Cirielli del 2005, una legge clemente verso la corruzione, mite sino ai limiti dell'indulgenzialismo per i rei incensurati (che tutte le statistiche peraltro dimostrano appartenere alle classi più agiate), ed invece escludente, discriminatoria ed antigarantista per i cosiddetti *outsider* sociali; proprio quell'idea di giustizia debole con i forti e forte con i deboli che andrebbe ribaltata in radice. Furono quelle norme, in particolare, a generare la situazione di oggi, incrementando drammaticamente il numero dei carcerati in nome della demagogia e della illusoria tolleranza zero, che prevedeva solo ed esclusivamente la centralità della pena detentiva quale strumento risolutorio dei casi di devianza sociale. Quella legge, che introduceva la figura del recidivo reiterato, destinatario di pene molto più lunghe a prescindere dalla gravità del reato, e la riduzione dei tempi di prescrizione non in relazione alla tipologia del reato, bensì in relazione al trascorso dell'imputato, con l'immediato effetto di una dura repressione dei comportamenti penali spesso legati a reati minori, era il manifesto ideologico di un preciso pensiero politico. È con questa tendenza che oggi si dovrebbe provare ad operare una vera cesura, che avremmo voluto molto più netta di quella di cui stiamo parlando; quella tendenza a rimuovere dalla società i rei, i diversi, gli ultimi, senza che peraltro questo autoritarismo, sperimentato in questi anni con un sistema di norme tese a criminalizzare comportamenti sociali diffusi (si pensi ancora una volta all'ossessione securitaria della legge Fini-Giovanardi in materia di droghe), sia riuscito minimamente ad intervenire sulla prevenzione o, ad esempio, sul contrasto alle mafie che gestiscono il narcotraffico. In Italia oggi i detenuti hanno già superato le 60.000 unità. Questo numero è molto più alto di quanto il sistema penitenziario possa reggere. Nelle nostre carceri si vive una condizione disumana e contro ogni dettato costituzionale, ci si ammala e si muore. Suicidi e atti di autolesionismo sono aumentati a dismisura, e non solo in regime di carcere duro. Un Paese civile non può più accettare una così profonda cancellazione dello Stato di diritto. È per questo che votiamo questo decreto, perché lo consideriamo appunto un passo avanti, perché inverte la tendenza di questi anni, perché il problema delle carceri e del sistema delle pene non è una questione che riguarda solo la popolazione detenuta e solo gli addetti ai lavori, perché bisogna rompere l'idea malata di un regime garantista per i garantiti e giustizialista per i socialmente giustiziati, perché sul rispetto dei diritti umani,

È una posizione che abbiamo già manifestato più volte in Commissione. Adesso veniamo qui a rendere una dichiarazione finale su qualcosa che noi riteniamo essere assolutamente scellerato. scellerato. La volontà del Governo di affrontare un problema come quello del sovraffollamento nelle carceri con questi rimedi non ci può trovare che all'opposizione. Sono solo delle soluzioni provvisorie, temporanee, ma che stanno provocando e provocheranno non poche ripercussioni anche sul nostro vivere civile.

Quello che mi sorprende è ciò che la stessa Commissione ha per certi versi ulteriormente appesantito.

questa mattina, tutti noi siamo stati responsabili nel prendere in considerazione la posizione dei recidivi. Ricordiamo che nel testo originario del Governo, purtroppo - dico veramente purtroppo - erano state eliminate delle previsioni dei limiti di accesso a questi benefici proprio ai recidivi. Fortunatamente - lo ripeto - l'esito dell'esame di questa mattina ha portato in una direzione diversa. Però mi sorprende pensare che il Governo, per risolvere un problema come quello del sovraffollamento delle carceri, abbia pensato ancora di beneficiare i recidivi, che - ricordiamo - sono tali perché hanno una propensione al reato e alla vita delinquenziale.

E quindi liberazione anticipata, sospensione della pena, detenzione domiciliare. Ma non ho ancora finito. Anche su un altro punto ritengo che sia importante soffermarci:

senza avere nulla nei confronti dei tossicodipendenti o degli utilizzatori di sostanze psicotrope, che sicuramente versano in una situazione particolare. Però la formulazione originaria della norma del decreto‑legge

I lavori di pubblica utilità sono veramente importanti, sono un modo di rieducare il condannato, però devono essere un qualcosa che si aggiunge, e non che si sostituisce, alla pena.

Noi della Lega Nord da tempo insistiamo sul fatto che l'unica maniera per risolvere il problema del sovraffollamento nelle carceri è di fare nuove strutture penitenziarie ed avere la possibilità di dare nuovi posti. C'era un piano carceri in opera. Ma non solo questo, ci sono dati molto importanti. Anche noi della Lega Nord abbiamo sempre sostenuto e continuiamo a ricordare a questo Governo e a voi tutti che all'interno delle nostre carceri, dove oggi sono presenti quasi 66.000 detenuti,

non si determina la misura delle carceri in base al numero dei criminali, ma il numero dei criminali dalla misura delle carceri. È questo forse che vogliamo?

ma se adesso adottiamo questi provvedimenti pur non avendole nemmeno iniziate, significa che stiamo affrontando falsamente un problema senza nemmeno conoscerlo, perché si dovevano fare le indagini conoscitive!

in cui sa a quale pena va incontro, il delinquente potrà essere dissuaso. Il nostro voto penso sia abbastanza chiaro. Il Gruppo Lega Nord esprime convintamente il suo dissenso.

abbiamo condiviso l'iniziativa del Governo, che si è aggiunta ad un'analoga iniziativa, più organica - per la verità - approvata dalla Camera dei deputati,

che certo non nasce oggi, ma che nei mesi e nelle settimane scorse ha raggiunto livelli non più accettabili. Un Paese civile, un grande Paese, non può tollerare di avere un sistema carcerario incapace di garantire il recupero del reo a una vita degna di essere vissuta. Certo, chi paragona le persone alle scimmie probabilmente fa fatica a capire questi principi di civiltà. *(Applausi

Per contro, l'opinione pubblica non è certo meno esigente nei confronti della necessità di salvaguardare un clima sociale di sicurezza e di lotta alla piccola e grande criminalità, a cui dobbiamo prestare la massima attenzione e a cui tendono anche gli emendamenti e i subemendamenti introdotti in Aula anche per raccogliere le preoccupazioni ed i suggerimenti espressi dalle stesse opposizioni in questa sede. In ogni caso, bisognava dare risposte urgenti rispetto al sovraffollamento delle carceri,

rafforzando la concezione della pena come ammenda e riducendo progressivamente la detenzione in carcere come misura tipica per i reati più gravi, quando si è in presenza di comprovato allarme o pericolosità sociale e quando non sussistono, per ragioni soggettive del reo o per ben definite condizioni oggettive, altre possibilità rispetto alla privazione della libertà personale attraverso il carcere. Questa è una battaglia lunga, non conclusa, tutt'altro che facile, che è un tutt'uno con una civiltà giudiziaria che si fonda sulla presunzione di innocenza, sul processo giusto, sull'effettiva parità tra accusa e difesa, sull'efficacia della pena, sulla celerità dei processi, sulla certezza della pena e, in sintesi, sulla certezza del diritto. Quindi, il provvedimento in esame, opportunamente corretto a seguito della discussione generale (ispirato da princìpi ben diversi da quelli che in passato hanno portato a indulti e amnistie, che si sono tradotti solo in «porte girevoli» per le persone beneficiarie), avrà il nostro voto favorevole. Auspichiamo, che presto si possa riesaminare la materia nel suo complesso, per dare una risposta organica e duratura ad una domanda di civiltà non disgiunta dalla tutela di quel bene primario per la convivenza delle persone che è la loro sicurezza civile e sociale.

già anticipato quello che sinteticamente andrò ad esporre fra non molto e che è stato già ampiamente illustrato dai colleghi del mio Gruppo politico che ieri hanno avuto la possibilità di intervenire, ovvero una avversità al decreto‑legge, così come come è arrivato dal Ministero, per il fatto di essere arrivato. Mi spiego meglio. La denuncia che svolgiamo quotidianamente, da settimane, da mesi, da quando siamo entrati in questo Palazzo, Palazzo, inerisce alla decretazione d'urgenza, ovvero alle modalità con cui in questo Paese, non da oggi e non certo per responsabilità in questa legislatura dei Ministri, del Presidente del Consiglio e quant'altro, da decenni andiamo avanti. Lo sappiamo: la produzione legislativa in questo Paese fa riferimento sostanzialmente al Governo, essendo ormai il Parlamento ridotto a mero notaio

Questo è un aspetto che noi continuiamo a non accettare e a stigmatizzare, richiamando anche quello che viene detto dai colleghi del Senato,

di lavoro non consentono al Parlamento di lavorare bene, cioè di licenziare provvedimenti legislativi che siano oltre che veloci anche utili al nostro Paese. La cronaca delle ultime ventiquattrore - credo possiamo dirlo - ce ne dà una conferma clamorosa. Nella giornata di ieri

alle difficoltà con cui la stessa maggioranza ha tentato di licenziare alcuni emendamenti, sicuramente rilevanti, e all'impossibilità pratica di poter lavorare in maniera dignitosa e adeguata al ruolo

compresi i membri della Commissione giustizia, hanno avuto la disponibilità delle 64 pagine di emendamenti e ordini del giorno, che comprendevano non solo quelli già approvati in Commissione, quindi magari già noti, ma anche quelli presentati

ribadito anche ieri dal presidente Gasparri; persino il senatore Giovanardi ha fatto riferimento alle ristrettezze temporali e alle incapacità operative con cui si è costretti a lavorare. Che l'argomento sia delicato e si debba mettere mano alla situazione nelle carceri è un qualcosa su cui è inutile insistere, e a noi non piace usare la retorica,

vergognato più volte del mio essere italiano di fronte alle disumanità a cui costringiamo i detenuti nel vivere nelle nostre carceri. Quindi, il problema

ci sembra un qualcosa da sottolineare e che giustifica il nostro voto contrario al decreto-legge nella sua interezza. Inoltre, ci fa ricordare tutte le perplessità che sin dall'inizio abbiamo manifestato con riferimento alla proroga della figura del Commissario straordinario. Anche in tal caso non abbiamo affatto condiviso la scelta che ci è stata proposta, se non quasi imposta, dal Ministero.

con riferimento alla presunta mancata copertura in relazione a un emendamento, proposto da una senatrice del Gruppo del Partito Democratico, volto a migliorare le condizioni sanitarie dei detenuti. Anche in quel caso sotto gli occhi di tutti si è palesata la frettolosità e la superficialità inevitabile con cui si è stati costretti ad affrontare un argomento così delicato. Quindi, riassumendo e condividendo nel merito la necessità di un intervento

alla luce alcune necessità di interlocuzione tra il Parlamento e il Governo, ed è venuta fuori una normativa che incide su alcune fondamentali questioni. questioni. Abbiamo detto che era meglio la detenzione domiciliare. Abbiamo disciplinato come tener conto della liberazione anticipata, che i tribunali di sorveglianza non avevano concesso, nonostante un periodo pregresso di carcerazione.

non solo io, ma tutti, ci siamo ispirati ad alcuni principi fondamentali. Il sistema penale si basa su un processo che sia assistito dalle garanzie della difesa e che sia accompagnato da una pena equa. L'equità della pena sta nella previsione astratta della legge, ma anche nel modo in cui la irroga il giudice, perché solo una pena equa può far avvertire al condannato la giustezza della sanzione e può consentire quello che la nostra Costituzione - e non solo la nostra tradizione giudaico‑cristiana - ci ha imposto: credere nella possibilità delle redenzione e di recuperare dopo aver sbagliato. Se così non fosse, dovremmo allora accettare ancora la pena di morte. Se l'abbiamo abolita, è perché ancora crediamo nella possibilità della redenzione e nel fatto che chi sbaglia deve pagare, ma deve pagare con un pena certa, signora Ministro, una pena che sia irrogata ed espiata, e deve esserci una differenziazione tra coloro che sbagliano la prima volta e quelli che sono criminali incalliti, quelli che sono recidivi specifici reiterati. È per questo che abbiamo creato una corretta diversificazione. Perché, vede, noi abbiamo caricato i tribunali di sorveglianza e i giudici dell'esecuzione di una serie di compiti: corretto. Però, signora siamo certi che questa riforma avrà attuazione? Lei sa che oggi in Commissione giustizia abbiamo chiesto una proroga della riforma delle circoscrizioni Lei sa meglio di me che, nelle occasioni in cui ci siamo incontrati, non ho mai fatto una questione di campanile. Mi interessa la funzionalità del sistema,

la soddisfazione dei diritti a poveri cristi, a chi non ha la possibilità di un avvocato e non ha la possibilità di attendere anni. Allora in questa vicenda dobbiamo garantire giudici di sorveglianza che immediatamente applichino le norme che abbiamo approvato e giudici dell'esecuzione che siano attenti a valutare quegli aspetti umani di cui abbiamo tenuto conto nella valutazione dei tossicodipendenti e di coloro che sono affetti da una certa situazione di malattia e di disagio.

Noi dobbiamo punire, ma punire nella certezza che, attraverso la sanzione penale, attraverso l'aiuto che lo Stato può dare

di fare una riflessione perché il sistema possa rispondere finalmente alle esigenze di giustizia. Presidente, colleghi, signora Ministro, è un primo passo, un passo nuovo, anche coraggioso. Naturalmente, signora Ministro, altri ne dobbiamo compiere, la strada è ancora lunga. Non si parte, finalmente, a valle, dall'indulto e dall'amnistia: con questo decreto si tenta di spostarci un po' più a monte. La condizione carceraria è difficilissima. Molti colleghi lo hanno spiegato bene: più di 65.000 persone

Si apre una strada nuova: arresti domiciliari, sospensione della pena, affidamento ai servizi, liberazione anticipata, lavoro volontario e gratuito, maggiore tutela e possibilità di cura per i tossicodipendenti. Nessun automatismo, colleghi, ma proprio nessuno. Quando il magistrato deve valutare gli arresti domiciliari, il primo criterio indicato nel decreto è tutelare le esigenze delle vittime del reato, e sono esclusi i reati più gravi: nessuna indulgenza da quest'Aula per i reati mafiosi; per i 41-*bis* nessuna opportunità, le porte sbattute in faccia; così per i reati che riguardano gli incendi boschivi, lo *stalking* e il maltrattamento dei minori, i furti gravi, i recidivi gravissimi, quelli reiterati e specifici. Per questo si sono volute calibrare due dimensioni molto importanti: trattamento e rieducazione, con una gamma articolata di esecuzione della pena, da un lato, sicurezza e rispetto per le vittime del reato,

padre esercente la potestà di prole di età inferiore ai dieci anni con lui convivente quando la madre sia deceduta o altrimenti impossibilitata a dare assistenza alla prole; persone in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; persona di età superiore ai sessant'anni, se inabile anche parzialmente; persona di età minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

discorso sui circuiti carcerari. Sì, signora Ministro, abbiamo voluto inserire un emendamento nel decreto in esame perché crediamo che la pena debba essere differenziata. Dobbiamo avere una gamma di opportunità di detenzione che non sia quella del classico polo cui concentrare tutti i detenuti: i megapoli, importanti ma insufficienti. Ci sono piccole strutture, sebbene organizzate, moderne e avanzate, dove si possono fare sperimentazioni, dove la differenziazione può diventare concretezza e realtà. Vi sono altri provvedimenti, Ministro, su cui dobbiamo intervenire: mi riferisco al personale, dai giudici di sorveglianza agli operatori, dagli educatori agli assistenti sociali e alla Polizia penitenziaria. Bisogna fare attenzione, perché, quando si scende troppo al di sotto degli organici, quando per loro diventa dura, tutte le riforme rischiano di fallire: le buone riforme devono avere risorse umane pronte, preparate e ben retribuite. Rimangono aperte alcune sfide, Ministro, e voglio solo accennare ad una che mi sta particolarmente a cuore: per spostarci veramente a monte e non rimanere a metà strada dobbiamo avere il coraggio di fare una riflessione moderna e avanzata sui tre gradi di giudizio. Forse è giunto il momento non magari di ridurli ma di articolarli bene,

abbiamo bisogno di lavorare di più, abbiamo bisogno di un Parlamento che abbia un'interlocuzione moderna con il Governo e di un Governo che abbia un'interlocuzione altrettanto costante con il Parlamento. Confidiamo nella sua responsabilità, Ministro, e quando parliamo di Commissario per la riorganizzazione dell'edilizia per quanto riguarda le carceri sappiamo che tocchiamo un punto delicato, sappiamo che lì, spesso, si sono annidati la corruzione e l'aggiramento delle norme di trasparenza e di legalità. Lei, Ministro, ha una storia nobile; sa anche, attraverso la sua storia, come controllare: eserciti tutti i suoi poteri e metta a frutto la sua esperienza per dimostrare che la scelta del Commissario è una scelta di modernità e non è la classica scorciatoia dell'«Italietta». Ministro, è un passo su cui noi vigileremo. Vorremmo interloquire con lei, ecco perché ci saranno delle relazioni che terranno informato il Parlamento, dal momento che, Ministro, vorremmo fare insieme tanti altri passi veri di riforma, per cui finalmente il trattamento e la rieducazione, la sicurezza e il rispetto delle vittime del reato diventino una realtà, un fatto di civiltà, attraverso cui possiamo guardare al nostro Paese e dire a Strasburgo che non ci faremo più punire perché siamo seri e perché la nostra civiltà giuridica ce lo impone.

internati, che vanno parificati ovviamente ai detenuti. Infatti queste misure si applicano, oltre che ai destinatari di una sanzione penale criminale, anche ai destinatari di una misura di sicurezza. proposta di coordinamento attiene all'articolo 4, come modificato dall'emendamento 4.8. Vi era in premessa un'espressione del tutto ultronea, «Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente». Si è pensato di sopprimerla proprio per la ridondanza e l'inutilità di un'espressione che è implicata ovviamente dall'esistenza di un panorama normativo al quale le leggi intervenute devono fare riferimento.

alla violenza sessuale, alla violenza di gruppo, alla violenza sessuale sui minori, mi chiedo allora: visto che in questa Aula, con tante colleghe e colleghi,

denunciato, non dirò in realtà quel che penso veramente di questa sentenza, ma ci tenevo a informare in quest'Aula, perché ne siano a conoscenza tutti. Credo che questa sia

recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti***

onorevoli senatori, il presente decreto-legge è il primo provvedimento del Governo che, anche se in modo parziale e nei limiti delle risorse disponibili, interviene al fine di promuovere l'occupazione, in particolare quella giovanile, in linea con le politiche assunte a livello europeo. Oltre alle suddette misure, il decreto reca disposizioni sulla coesione sociale e in materia di imposta sul valore aggiunto, che saranno illustrate dal relatore Sciascia, io mi occuperò della parte lavoristica. Il provvedimento si inserisce in una situazione di grave e prolungata difficoltà congiunturale ed in un contesto contrassegnato da una profonda crisi economica... *(Forte brusìo)*. PRESIDENTE. Colleghi, scusate, ma la relatrice non riesce a sovrastare con la sua voce il brusìo,

Dicevo che il provvedimento si inserisce in una situazione di grave e prolungata difficoltà congiunturale e in un contesto contrassegnato da una profonda crisi socio-economica, che investe il nostro Paese ormai da diversi anni, i cui riflessi sul mondo del lavoro e sui livelli occupazionali richiedono richiedono interventi strutturali e di sistema. Nei primi tre mesi dell'anno - come confermato dalla Banca d'Italia - il prodotto interno lordo è stato inferiore dell'8,7 al massimo ciclico raggiunto nel 1° trimestre del 2008. Nell'intero quinquennio 2008-2012, la caduta dell'attività in Italia è stata la più marcata tra i maggiori Paesi dell'Unione europea. La situazione del mercato del lavoro italiano

La situazione del mercato del lavoro italiano si è però notevolmente aggravata dalla seconda metà del 2011. In concomitanza con la crisi dei debiti sovrani, la modesta ripresa seguita alla recessione mondiale del 2008-2009 si è arrestata e tramutata in una nuova pesante recessione, che ha frenato la domanda di lavoro espressa dalle imprese. La disoccupazione giovanile è una grande emergenza da risolvere nel nostro Paese, se vogliamo garantire all'Italia un futuro di ripresa e nuovo sviluppo. L'incidenza della disoccupazione è, infatti, maggiore per le classi di età più giovani (in particolare quelli con meno di venticinque anni). In questo contesto, il provvedimento del Governo rappresenta un passo importante, anche rispetto al passato, nella lotta alla disoccupazione. Ciò nonostante, ci auguriamo che sia solo il primo passo di un lungo percorso. È infatti necessario proseguire con provvedimenti ancora più coraggiosi, reperendo nuove risorse che, oltre agli incentivi per le assunzioni, mirino a riformare il sistema creando le condizioni per promuovere nuovi investimenti. Restano da sciogliere nodi importanti, come il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e della piccola mobilità per le piccole imprese, la questione degli esodati e la questione del blocco dell'aumento dell'IVA nel settore sociosanitario. Si tratta di vere e proprie emergenze sociali. Insomma, vanno assunti altri provvedimenti, onerosi e strutturali, che le risorse disponibili in questo provvedimento non permettono di affrontare. Pur avendo approvato il decreto-legge senza modifiche sostanziali, le Commissioni riunite finanze e lavoro hanno apportato miglioramenti al testo originario, ovviamente limitati nella loro portata dal fatto che non sono state stanziate ulteriori risorse. In questa relazione darò conto di una breve sintesi delle misure previste dal decreto-legge e della loro portata innovativa e delle modifiche approvate dalle Commissioni riunite. L'articolo 1 introduce una misura di incentivo temporaneo, in favore dei datori di lavoro, per la stipulazione di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con soggetti di età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, che diano luogo ad un incremento occupazionale netto, nonché per le trasformazioni di contratti di lavoro dipendente da tempo determinato a tempo indeterminato, accompagnate da ulteriori assunzioni ad incremento. Si tratta di un primo intervento che va nella giusta direzione per combattere la disoccupazione giovanile, che nel nostro Paese raggiunge ormai quasi il 40 L'intervento è finalizzato ad incentivare la creazione di lavoro a tempo indeterminato, l'autoimprenditorialità e l'impresa sociale e ad avvicinare i giovani che non studiano e non lavorano (i famosi al lavoro attraverso tirocini, nonché a contrastare la povertà estrema. Emendamenti approvati dalle Commissioni riunite comportano lo snellimento e il chiarimento delle procedure

l'introduzione del termine temporale di un mese entro il quale la suddetta trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato deve essere accompagnata da un'ulteriore assunzione ad incremento e la previsione che l'incentivo sia oggetto di monitoraggio e di valutazione. Vorrei segnalare poi che sull'articolo 1 sono stati presentati diversi emendamenti, non accolti dalle Commissioni riunite, finalizzati ad innalzare fino a trentacinque anni l'età dei giovani per la cui assunzione sono previsti incentivi per i datori di lavoro, e che lo stesso tema è stato presente nel dibattito pubblico. L'innalzamento sembrerebbe però non possibile, in quanto in contrasto con quanto previsto dal regolamento CE n. 800 del 2008, alla base delle disposizioni che regolano l'erogazione dell'incentivo. L'articolo 2, nei commi da 1 a 9, mira a realizzare una disciplina dell'apprendistato più omogenea sull'intero territorio nazionale. Naturalmente è necessario che i principi previsti siano tradotti al più presto in disposizioni concrete e direttamente applicabili mediante le linee guida da individuare in Conferenza Stato-Regioni. L'emendamento 2.500, approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone la soppressione della disposizione per cui, laddove le Regioni e le Province autonome non abbiano adottato specifiche regolamentazioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, trova applicazione la normativa statale in materia e della disposizione per cui, anche per i tirocini instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, sia corrisposta al tirocinante l'indennità di partecipazione. Si ricorda che la soppressione del comma 4 è stata posta come condizione nel parere non ostativo espresso dalla 1ª Commissione del Senato sul decreto-legge in esame. propone l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un fondo straordinario, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», con una dotazione pari a 1 milione di euro per il 2014, destinato alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento, rivolti ai giovani fino a ventinove anni di età,

L'articolo 2, nei commi 10-14, incentiva le attività di tirocinio curriculare svolte dagli studenti universitari nell'anno accademico 2013‑2014. Con l'emendamento 2.24 è stata modificata la norma che prevede la possibilità di assegnare allo studente gli incentivi quale cofinanziamento, per metà, del rimborso spese corrisposto da altro soggetto pubblico. Con l'emendamento citato, nella nozione di «rimborso» rientra anche il beneficio o la facilitazione non monetaria, solo per i tirocini all'estero. L'articolo 3 reca misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno. Gli emendamenti 3.2 e 3.3, approvati nel corso dell'esame in sede referente, propongono di esplicitare che i progetti summenzionati, relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno, sono promossi, oltre che dai giovani e dai soggetti delle categorie svantaggiate, anche dai soggetti delle categorie molto svantaggiate e che i medesimi progetti devono fare particolare riferimento ai beni immobili confiscati ai sensi della legislazione antimafia. L'emendamento 3.4 (testo 2), anch'esso approvato nel corso dell'esame, pone un criterio di priorità - in favore di progetti o imprese in grado di contare su un'azione di accompagnamento e tutoraggio da parte di altra impresa già operante da tempo, con successo, in altro luogo e nella medesima attività nell'ambito degli stanziamenti summenzionati relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, ai progetti inerenti all'infrastrutturazione sociale ed alla valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno. L'articolo 4 reca misure dirette ad accelerare le procedure di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali europei e di rimodulazione del Piano di azione coesione. L'articolo 5 istituisce, in via sperimentale, una struttura di missione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente compiti di promozione, indirizzo, coordinamento, definizione di linee guida predisposizione di rapporti, con riferimento all'attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, del programma comunitario «Garanzia per i giovani» (*Youth Guarantee*), alla ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale e, in particolare, degli ammortizzatori sociali in deroga. 2) e 5.500 (testo corretto), anch'essi approvati, propongono alcune modifiche ed integrazioni alle norme di individuazione dei compiti della nuova struttura di missione. In particolare, l'emendamento 5.500 (testo corretto) dei relatori propone che la definizione dei criteri per l'impiego delle risorse economiche, relative alle politiche attive del lavoro, sia operata anche in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. L'articolo 6 intende favorire un raccordo organico tra i percorsi degli istituti statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. L'articolo 7 reca modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, attenuando alcuni vincoli normativi relativi ai contratti di lavoro più flessibili. che deve intercorrere tra due contratti a tempo determinato stipulati tra un'impresa e uno stesso lavoratore (da novanta a venti giorni per i contratti con durata iniziale oltre i sei mesi e da sessanta a dieci giorni per quelli sotto i sei mesi); si elimina il divieto di prorogare un contratto a tempo determinato stipulato senza specificarne la causale e si estende la possibilità, per i contratti collettivi nazionali o aziendali, di individuare situazioni in cui non è richiesto di specificare tale causale; si amplia la possibilità di ricorrere al lavoro intermittente, al lavoro accessorio e ai contratti di collaborazione coordinata; si consente al datore di lavoro di riassumere con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, mirante al conseguimento della qualifica professionale valida ai fini contrattuali, il lavoratore che abbia conseguito una qualifica o diploma professionale nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato, prolungando così la fruizione dei relativi incentivi contributivi. L'emendamento 7.39, anch'esso approvato, propone l'inserimento di una modifica con la quale si consente, senza la condizione della sussistenza di un interesse, il distacco temporaneo di lavoratori nell'ambito di imprese che abbiano sottoscritto un medesimo contratto di rete di impresa e si prevede che quest'ultimo possa definire le regole per ipotesi di codatorialità di dipendenti da parte delle imprese sottoscrittrici. Viene anche modificata la disciplina dell'istituto del lavoro intermittente. L'emendamento 7.45, approvato anch'esso, propone di esplicitare che i limiti di impiego si riferiscono a ciascun datore di lavoro. Sul lavoro a progetto, l'emendamento 7.70 propone di chiarire l'ambito di applicazione della norma che fa salvo il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. L'emendamento in esame propone di chiarire che tale norma si riferisca alle attività di vendita diretta di beni e alle attività di vendita di servizi, realizzate attraverso *call center outbound*, specificando, dunque, che l'aggettivo «diretta» si riferisce esclusivamente alla vendita di beni e non anche alla vendita di servizi. L'articolo 8 istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive, per favorire un migliore incontro tra domanda e offerta dì lavoro in termini di qualifiche e capacità, stimolando così occupazione, produttività e crescita. L'emendamento 8.500 (testo corretto), approvato nel corso dell'esame in sede referente, propone l'inserimento di altri soggetti nell'elenco di quelli che concorrono alla costituzione della banca dati. Sull'articolo 9, che tra l'altro reca alcune norme relative ai soggetti extracomunitari, merita di essere menzionato l'emendamento 9.32, approvato anch'esso, che propone di ampliare l'ambito dei soggetti extracomunitari che, al termine di determinati corsi di studio e alla scadenza del relativo permesso di soggiorno (per (per motivi di studio), hanno diritto di essere iscritti nell'elenco anagrafico dei centri per l'impiego, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero di chiedere, in presenza dei requisiti stabiliti dalla relativa disciplina, la conversione del permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nella disciplina vigente, tali possibilità sono riconosciute al soggetto extracomunitario che abbia conseguito in Italia un dottorato o un *master* universitario di secondo livello. L'emendamento 9.32 in esame propone un'estensione ai casi di conseguimento (in Italia) di una laurea triennale o di una laurea specialistica. L'articolo 10 reca alcune disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali, mentre l'articolo 11, in alcuni commi, disciplina le attività di rimozione delle macerie e terra miste ad amianto nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nonché in quelle interessate dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 e al comma 17 autorizza il Ministero dei beni e le attività culturali ad erogare tutti i fondi residui del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di fronteggiarne lo stato di crisi e di salvaguardare i lavoratori. Concludendo, signora Presidente, sono urgenti e non più differibili le finalità del provvedimento in esame, quali l'accelerazione della creazione di posti lavoro a tempo determinato e indeterminato (con particolare riferimento ai giovani e ai disoccupati), l'anticipo della cosiddetta garanzia giovani la politica europea che partirà dal 1° gennaio 2014), gli interventi in materia previdenziale e di politiche sociali, il rafforzamento delle tutele per i lavoratori e gli interventi per le imprese. Ciò nonostante, l'urgenza di affrontare una congiuntura economica così complessa, e per più aspetti drammatica, dovrebbe indurre il Governo e lo stesso legislatore ad adottare scelte più nette e incisive al fine di rilanciare le dinamiche occupazionali in tutti i settori produttivi;

Signora Presidente, signori del Governo, onorevoli senatori, il provvedimento in esame, già ampiamente illustrato dalla collega Gatti soprattutto per la parte (preponderante) concernente le modifiche alla disciplina dei rapporti di lavoro, cioè gli articoli da 1 a 10, dispone anche (agli articoli 11 e 12) nuove disposizioni in materia fiscale che andremo ad esaminare in modo estremamente sintetico. Cardine delle disposizioni fiscali è il rinvio dell'aumento dell'aliquota IVA cosiddetta normale, dall'attuale 21 per

La legge di stabilità per il 2013 ha messo un punto fermo, prevedendo unicamente l'aumento di un punto dell'aliquota normale, con conferma quindi sia della ridotta che dell'agevolata. alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 11, viene abrogata la disposizione che prevedeva l'inapplicabilità dell'aumento ove, entro il 30 giugno 2013, fossero entrati in vigore provvedimenti atti a ridurre sia le spese che i regimi di esclusione o limitazione delle basi imponibili sia per le imposte dirette che per l'IVA, di entità tale da comportare riduzioni dell'indebitamento netto non inferiori a 6.560 milioni di euro. Secondo la scheda tecnica allegata al provvedimento, il differimento dell'aumento d'aliquota al 1° ottobre 2013 comporta un onere finanziario di ben 1.059 milioni. Peraltro in sede delle audizioni effettuate sull'argomento presso le Commissioni, è stato affermato, tra l'altro e quasi all'unanimità, che tale aumento potrebbe determinare un decremento degli acquisti, proprio per il conseguente aumento dei prezzi determinato da un'IVA al 22 per cento, aumento che avrebbe una

per il trasferimento alla Grecia, da parte degli Stati firmatari, dei profitti derivanti dai titoli di Stato ellenici in carico all'Eurosistema nonché di quelli in carico alle Banche centrali nazionali, ivi compresa la Banca d'Italia. La quota di utili di competenza del nostro Paese è di 4,1 milioni di euro che, con complesse operazioni contabili, saranno accreditate alla Grecia. Al comma 5 si dà attuazione all'accordo del maggio 2011, secondo cui il nostro Paese deve contribuire per 26,1 milioni di euro al finanziamento della messa in sicurezza (il cosiddetto sarcofago) del reattore nucleare di Chernobyl. Il versamento sarà però solo di 25,1 milioni, per la presenza di un residuo attivo di 1 milione, e sarà così scadenzato: 2 milioni nel 2013; 5,775 milioni in ulteriori 4 rate annuali di pari importo. Al comma 6 viene corretto (con un onere di 17.000 euro) l'errata contabilizzazione del nostro contributo alla ricostruzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo. Ai commi 7 e 8 vengono riscritte le disposizioni per la detassazione di plusvalenze e sopravvenienze attive determinate da indennizzi, risarcimenti o contributi di natura sia pubblica che privata in favore delle imprese danneggiate dal sisma del maggio 2012, ivi compresi quindi - e questa è la novità - i lavoratori autonomi. Ai presidenti delle Regioni interessate è attribuito il compito di procedere agli opportuni controlli.

dalle conseguenti necessarie demolizioni e, infine, dalla tromba d'aria del maggio 2013. Tali operazioni saranno effettuate dai gestori dei pubblici servizi.

nonché le Province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall'anno 2014, potranno maggiorare l'aliquota base dell'addizionale regionale

dell'anticipazione di liquidità già erogata dallo Stato sia per debiti commerciali, che per quelli del Servizio sanitario nazionale. Con i commi da 13 a 16, con una serie di complesse norme viene delineata la procedura per la riqualificazione e la definizione dei piani di rientro per il sistema di mobilità su rotaie della Regione Campania. Viene disposta l'erogazione di prestiti di rilevante importo. Per l'ammortamento dei prestiti di cui si è detto

comma 17 viene autorizzata per il 2013 l'erogazione a favore delle fondazioni lirico sinfoniche di tutti i residui del Fondo unico per lo spettacolo (FUS). I commi 18, 19 e 20 contengono disposizioni atte a compensare le perdite di gettito derivanti dalle posposizioni dell'aumento dell'aliquota IVA. In particolare, si aumenta dal 99 al 100 per cento l'acconto IRPEF, a partire già dal corrente anno (con conguaglio sulla rata di novembre per il solo 2013), e si aumenta dal 100 al 101 per cento l'acconto IRES (Imposta sul reddito delle società). Anche in questo caso si opererà il conguaglio sulla seconda rata. A differenza dell'aumento di cui in precedenza (quello IRPEF disposto in via continuativa) l'aumento IRES opererà unicamente per il solo periodo d'imposta in corso al 31 2013. Gli aumenti già indicati, per esplicita disposizione del decreto legislativo n. 442 del 15 dicembre 1997 hanno effetto anche per l'IRAP, i cui acconti risultano così variati: per le persone fisiche e le società di persone dal 99 al 100 per cento, per i soggetti IRES dal 100 al 101 per cento. In materia di acconti è opportuno precisare che gli stessi vengono così determinati: con il metodo storico, cioè prendendo a base quanto pagato nell'anno precedente (o nel periodo d'imposta precedente) e con il metodo previsionale, cioè determinando l'acconto sulla base di una stima

comma 21 si dispone che per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo gli istituti di credito dovranno versare un acconto pari al 110 delle ritenute dagli stessi operate sugli interessi maturati su conti correnti ed i depositi. Con i commi 22 e 23 viene introdotta, a partire dal 1° gennaio 2014, un'imposta di consumo del 58,5 per cento sui prodotti «contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo». In pratica, sono colpiti dalla nuova imposta le cosiddette sigarette elettroniche. Vengono altresì disposte una serie di norme che introducono (sempre dal 2014) disposizioni per l'apertura e la gestione di esercizi per la vendita di tali prodotti. Tale normativa, particolarmente articolata, in pratica ricalca quella oggi in vigore per la vendita dei tabacchi con tutti i controlli e le sanzioni disposti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si dispone, infine, che il Ministero della salute promuoverà le opportune iniziative in materia per la tutela della salute. tutta una serie di disposizioni per assicurare la copertura finanziaria delle operazioni evidenziate. *(Applausi

Devo, in via preliminare, dichiarare cosa tristemente non mi sorprende, ovvero il fatto che siamo di fronte all'ennesimo decreto-legge *omnibus,* ampio contenitore che questo, come ogni precedente Governo, riempie in maniera assolutamente eterogenea con provvedimenti d'emergenza veri, indotti o presunti. Premesso ciò, la prima sorpresa (articolo 11, comma 5) riguarda tutti coloro che ancora parlano di nucleare sicuro. Di sicuro c'è il fatto che, laddove in una centrale nucleare qualcosa non vada per il verso giusto, le conseguenze, anche di carattere economico, le pagheranno le (due, tre, dieci?) generazioni successive. Infatti, l'Italia contribuirà con 25 milioni di euro all'ennesima e (vorrei poter dire ultima, ma sarebbe eccesso di ottimismo) ricostruzione del sarcofago di Chernobyl. Preciso, perché mi sembra giusto farlo per chi ascolta, che si tratta esattamente della stessa Chernobyl dove accadde quel piccolo "incidente" nel lontano 1986. Altra sorpresa (articolo 11, commi 12 e 15) è dedicata ai cittadini di Trento e Bolzano, nonché a quelli delle Regioni a Statuto speciale e della Regione Campania, i quali vedranno lievitare le proprie addizionali regionali IRPEF (e, nel caso della Campania, anche dell'IRAP) per far fronte ad una serie di debiti delle rispettive Regioni, del Servizio sanitario nazionale e della pubblica amministrazione. In un momento congiunturale come 1'attuale sarà certamente una sorpresa gradita. Ma è passando ai commi dell'articolo 11 dal 18 al 20 che le sorprese si fanno più interessanti. Si tratta di quei commi nei quali si sancisce che, per far fronte alle risorse finanziarie richieste dal decreto, e mi riferisco in particolare allo slittamento dell'aumento dell'IVA, si fa ricorso ad un incremento di un punto percentuale degli acconti IRPEF, IRES e conseguentemente IRAP. Allora, colleghi, cerchiamo di intenderci: siamo nello stesso Paese in cui chiude un'azienda al minuto? Siamo nello stesso Paese che affronta un costante calo del potere d'acquisto dei cittadini ed un contemporaneo costante aumento dei disoccupati e dei poveri ? L'ISTAT parla di un 15,8 per cento di italiani in situazione di povertà, dei quali l'8 per cento in povertà assoluta. Siamo nello stesso Paese il cui Governo ha celebrato come un evento storico aver pagato parzialmente e in maniera dilazionata i debiti dello Stato alle imprese, dando finalmente a queste ultime un po' di respiro? Se siamo nello stesso Paese, allora questo provvedimento è l'equivalente del gioco delle tre carte: un gioco in cui, con una mano, lo Stato posticipa una imposta indiretta e, con l'altra, copre questa dilazione con un maggiore anticipo di una imposta diretta. Peccato che, stanti i dati congiunturali di cui tutti siamo a conoscenza e che ormai ripetiamo in quest'Aula in occasione di ogni provvedimento e fatto salvo un improbabile *boom* economico, tale maggiore anticipo viene calcolato su un imponibile inesistente e si trasformerà in massima parte in crediti d'imposta. Nelle scorse settimane il senatore Calderoli ha utilizzato il termine "furto di Stato". Io voglio essere più diplomatico e parlare di «prestito forzoso a tasso zero». A parte il fatto che ci si è rivolti alla banca sbagliata, forse potremmo chiederci a quanti cittadini e a quante imprese sarebbe concesso un tale privilegio. Andiamo oltre. Parlando del comma 22 dell'articolo 11, la sorpresa in questo caso non è tanto nell'aumento della tassazione sulle cosiddette sigarette elettroniche, quanto nella giustificazione che, nella relazione di accompagnamento si dà a tale aumento. Cito testualmente: «salvaguardia delle entrate erariali derivanti dal consumo dei tabacchi lavorati, in particolare delle sigarette, le quali subiscono l'effetto sostitutivo del consumo (...) di detti succedanei». Ma in questa frase la tutela della salute dov'è? Se ammettiamo che le sigarette elettroniche fanno diminuire il consumo di quei prodotti che recano la scritta «Nuoce gravemente alla salute», sarebbe auspicabile determinare in via preliminare e definitiva se questa circostanza possa ridurre la spesa sanitaria nazionale, e solo successivamente decidere se aumentare la tassazione o no. Se invece si determinasse che tali succedanei possono comunque arrecare danno alla salute, sarebbe una notizia da comunicare immediatamente ai cittadini, senza attendere gli esiti del futuro monitoraggio previsto dal comma 23. Le ultime sorprese fornisce l'articolo 12. Alla lettera *e)* scopriamo che uno dei pochi provvedimenti positivi attribuibili al precedente Governo, ovvero 1'istituzione di un fondo per l'esclusione dall'IRAP delle persone fisiche che esercitino attività commerciali, artigianali e professionali senza dipendenti e con limitati beni strumentali, viene sostanzialmente dissanguato per finanziare il provvedimento oggi Immagino che, in considerazione del fatto che tale fondo non sia mai stato effettivamente utilizzato, si sia pensato di svuotarlo definitivamente e di togliersi il pensiero. Del resto, c'era il rischio che portasse qualche beneficio all'economia. Infine, la lettera *f)* dell'articolo 12 ci regala la sorpresa più grande: il *premier* Letta si dimetterà. E lo dico chiedendo un po' di attenzione al Governo. Nel corso di un'intervista rilasciata il 5 maggio nel corso della trasmissione «Che tempo che fa» questi dichiarava (cito testualmente): «Io mi dimetto se dovremo fare dei tagli alla cultura, alla ricerca e all'università». Non mi ritengo un fine cultore della lingua italiana, ma quando leggo, alla lettera *f)* dell'articolo 12: «quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento ordinario delle Università», immagino che in qualche modo si parli di tagli all'università! Sono convinto che il *Premier*, che valuto un uomo di parola, ne trarrebbe le dovute conseguenze, ma invito questa Assemblea - e in particolare la maggioranza che questo *Premier* sostiene - a sottrarlo a un destino, che sicuramente è frutto di una svista, votando convintamente gli emendamenti del Gruppo del Movimento 5 Stelle volti a individuare fonti di finanziamento alternative. 890** Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli senatori, in merito al provvedimento oggi in discussione voglio esprimere alcune considerazioni di fondo, vista l'importanza delle tematiche in esso affrontate. Per quanto attiene alle misure sull'occupazione è da apprezzare lo sforzo governativo per gli incentivi alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e gli interventi straordinari per l'occupazione giovanile che consentiranno il coinvolgimento occupazionale di una numerosa platea di giovani che avranno la possibilità di sperimentare nuove forme di occasioni professionali anche in concomitanza degli studi. L'articolo 3 del decreto-legge n. 76 prevede inoltre una serie di azioni contro la povertà nel Mezzogiorno che sembrano tuttavia dettate, in parte, più dalla necessità di accelerare la spesa dei fondi europei che non da una programmazione strutturata effettuata di concerto con le Regioni. Alcune azioni contenute al comma 1 dello stesso articolo prevedono la possibilità della valorizzazione di beni pubblici nel Mezzogiorno ma non vengano opportunamente specificato modalità e tempistiche attuative. Il tema del recupero del patrimonio pubblico per favorire la nascita di nuove imprese giovanili ritengo sia un argomento sul quale bisognerà maggiormente impegnarsi nel futuro della legislatura prevedendo azioni immediate. Dobbiamo puntare a promuovere il recupero e la riconversione di siti industriali dismessi, anche sottratti alle organizzazioni criminali, e presenti negli agglomerati industriali sparsi sul territorio nazionale ed in particolare rivitalizzare aree e strutture che hanno beneficiato in passato di finanziamenti e contributi pubblici non andati a buon fine. A tal fine sarebbe opportuno elaborare azioni di promozione e recupero del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 63 della legge n. 448 del 1998 per convertire gli opifici industriali in incubatori di imprese da offrire in locazione gratuita, per un periodo massimo di cinque anni, in favore di nuove imprese costituite da giovani o soggetti svantaggiati che vogliono ripartire ma che mancano delle opportune facilitazioni. Voglio inoltre esprimere perplessità riguardo lo sconto contributivo ai giovani tra i 18 e 29 anni che si sovrappone con il trattamento contributivo del contratto di apprendistato. Il decreto, infatti, intervenendo sul piano formativo e sulla formazione di competenza regionale, conferma l'istituto dell'apprendistato quale canale privilegiato per l'accesso al mercato del lavoro dei giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Il contratto di apprendistato ha una finalità formativa, mentre l'incentivo di cui al decreto-legge in questione è diretto ad un mero inserimento occupazionale. Ciò detto, in un'ottica comparativa sul piano dei costi, molto probabilmente l'intervento del Governo rischia di

e se il concetto di primo rapporto, ovviamente di natura subordinata, possa incontrare un limite temporale nella prescrizione decennale. Sul piano letterale e in relazione a come è stato strutturato il nuovo comma 1-*bis*, sembrerebbe ragionevole ritenere che il limite dei dodici mesi si riferisca solo all'ipotesi legale di cui alla lettera Tale situazione renderebbe più ampio e facile il ricorso al co.co.pro, e aumenterebbe il rischio di elusione della stipula di contratti a tempo determinato. In chiusura, auspicando nuovamente l'elaborazione di nuovi e più incisivi strumenti di rilancio dei consumi anche attraverso la definitiva soluzione del blocco dell'aumento IVA - differito al 1° ottobre - e in relazione alle misure per contrastare la disoccupazione giovanile, concentriamo l'attenzione sull'obiettivo della nostra azione

E indicare una direzione di marcia è compito della politica, anche in questo tempo di grande disaffezione dei cittadini e delle cittadine. Penso che tutti noi in quest'Aula, al di là degli schieramenti, dobbiamo sentire la responsabilità di trovare soluzioni concrete ed infondere anche fiducia nel futuro. Perché la conversione in legge del decreto-legge n. 76 indica una direzione di marcia che deve necessariamente portare a politiche di sistema, come ho avuto anche l'onore di dire in occasione della discussione sulla fiducia al Governo Letta? Perché è la prima volta, nella complessità (ricordata da tutti) di questo provvedimento, che si mette al centro l'occupazione giovanile. Cito tre esempi di questo aspetto presenti nel decreto. La *ratio* del provvedimento è nell'articolo 1, in cui si prevedono incentivi alle aziende per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Aiutare le aziende in un momento di grave crisi economica e affrontare con energia la disoccupazione giovanile sono i due pilastri su cui si costruisce il futuro. In più in questo articolo, con la previsione di assunzioni di giovani a tempo indeterminato, si intende stabilizzare il lavoro in un Paese in cui, come testimoniano i dati OCSE, è precario il 52 per cento dei giovani sotto i 25 anni: il doppio rispetto al 2010. Il secondo esempio è dato dalla riprogrammazione di fondi europei nel Mezzogiorno terzo mi sta particolarmente a cuore. Nell'articolo 5 si stabiliscono misure per l'attuazione del programma europeo «Garanzia per i giovani» e per la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Si prevede a tal fine una struttura di missione presso il Ministero del lavoro. del lavoro. Questo non basta. È solo un primo passo. Dobbiamo andare verso la definizione di un sistema nazionale costituito da un'agenzia nazionale e da agenzie regionali. 19 Paesi su 28 (29 ora) in Europa dispongono di una struttura a rete o, più spesso, di un'agenzia nazionale dotata di strutture territoriali e, diversamente dal resto dell'Europa, in Italia, nel momento di massima crisi, si è investito poco in politiche attive. Riusciremo a costruire il futuro pure affrontando le emergenze, come questo Governo sta facendo, se realizzeremo servizi all'impiego efficienti e trasparenti, dove una ragazza o un ragazzo che cerca lavoro su tutto il territorio nazionale (perché uno dei problemi che abbiamo è che ci sono troppe asimmetrie territoriali) riuscirà a trovare accoglienza e risposte concrete di accompagnamento al lavoro. E questo vale anche per coloro che al momento non studiano e non lavorano perché scoraggiati. Queste non sono questioni tecniche, ma attengono alla necessità di creare sistemi trasparenti di accesso al lavoro.

Fondamentale è il raccordo tra le azioni che accrescono l'occupabilità dei soggetti e gli interventi a sostegno del reddito. In Europa è in atto un dibattito pubblico su come gli incentivi ai centri unici aumentano efficacia ed efficienza dell'azione in materia occupazionale. Il ruolo dei privati all'interno di un sistema nazionale del raccordo tra servizi pubblici all'impiego e programmazione formativa, che è sempre ricorrente nelle raccomandazioni del Consiglio europeo. Infine, pongo all'attenzione un tema che dovrà essere affrontato. In Commissione abbiamo sempre cercato di raccordare, naturalmente, le normative nazionali con l'azione della Conferenza Stato‑Regioni, ma credo che debba riflettere, monitorare e valutare, sia da parte dello Stato che da parte delle Regioni, il Titolo V della Costituzione in materia di lavoro. È complicato avere 20 forme di apprendistato

onorevoli colleghi, quanto è riuscito a fare il Governo sulla nota questione dell'IVA ha veramente dell'incredibile. Dopo le frementi proteste da parte delle associazioni di categoria, soprattutto del commercio, dei negozianti, delle imprese ha deciso di....non decidere! Ha semplicemente spostato il previsto aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA ad ottobre. Nel timore, infatti, di essere accusato di non intraprendere le istanze di chi in Italia produce ricchezza e lavoro val bene la pena di ricordarlo - l'Esecutivo si è preso 90 giorni di tempo per decidere. Tuttavia, mentre i rappresentanti del Governo spremeranno le loro meningi sotto l'ombrellone nel solleone agostano, c'è chi dovrà prepararsi, comunque finisca la triste saga dell'IVA, a rinunciare alle meritate vacanze per versare il prossimo novembre più acconti di tasse. E il merito è tutto vostro, Governo! In pratica, questo decreto sospende un aumento di tassazione con un altro aumento. Qualcuno ha paragonato questa mirabile idea al gioco delle tre carte: io ritengo che nemmeno David Copperfield sarebbe riuscito in una magia del genere. Una magia che farete pagare a quelle stesse aziende che un giorno affermata di voler sostenere, di voler rilanciare, per poi tassarle di più il giorno dopo. Anzi, questa volta siete riusciti addirittura a far meglio di quanto si potesse solo lontanamente immaginare: a novembre, infatti, l'aumento degli acconti IRPEF passerà dal 99 al 100 Il concetto è: prima paghi le tasse, dopo lavori. Forse. E i soggetti IRES addirittura, grazie alla vostra lungimirante idea, si troveranno a dover pagare l'acconto IRAP per un importo pari al cento del reddito non ancora prodotto! Oggi le aziende vivono una situazione economica nella quale non sono minimamente in grado di conoscere quali saranno i futuri andamenti del mercato nel quale operano, dove per "futuri" si intende uno spettro temporale di solo qualche mese. Forse però la cosa non vi è nota, se avete deciso perfino di superare l'attuale normativa, già di per sé assurda,

l'acconto delle tasse! È un vero raggiro nei confronti dei cittadini e delle imprese. Fa specie, poi, come abbiate deciso di affondare uno dei pochi settori aziendali che in questi mesi stava dando qualche segnale di positività. L'aumento, anzi, il raddoppio abbondante dell'imposta sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati e sui dispositivi meccanici ed elettronici (e non si capisce perché vengano tassati tali dispositivi), comunemente note comunemente note come "sigarette elettroniche", mette infatti al muro un settore che più di altri, in un momento di profonda crisi, stava dando delle possibilità di lavoro ai disoccupati. Il vostro è un vero colpo di mano: senza alcuna consultazione con i produttori state minacciando il comparto, con il rischio chiusura di almeno il 60-70 per cento dei punti vendita che - e questo è ancora più grave - porterebbe a perdere più di 3.000 posti di lavoro. Non era facile, ma ci siete riusciti! Complimenti, Governo! Non c'è quindi alcuna prospettiva di riforma strutturale in questo documento. E non potrebbe essere altrimenti, del resto: avete deciso di rinviare e rinviare, senza mai davvero adottare riforme strutturali e durature. Ci sarebbe quella, invero, dei costi *standard* (visto che tutti dicono che non ci sono soldi e la coperta è corta, ci sarebbe appunto questa riforma), opportunamente tralasciata dal Governo Monti e anche da voi oggi messa nel dimenticatoio. Ma volete mettere risparmiare risorse pubbliche facendo pagare a tutte le sanità regionali lo stesso prezzo per le siringhe con un aumento degli acconti delle imposte sui redditi d'impresa? Non sia mai che invece di agire, come sempre, sul lato della maggiorazione delle entrate tributarie, questo Governo decida di tagliare i rami secchi della spesa pubblica! Gli unici provvedimenti a favore di qualcuno, come al solito, li avete predisposti per i soliti noti. interessante osservare, infatti, la possibilità che concedete alla sola Regione Campania di poter dirottare risorse fresche per saldare i propri buchi in materia di trasporto regionale ferroviario: un atteggiamento certamente meritocratico verso chi ha sempre rispettato le regole, verso chi ha gestito con oculatezza le risorse pubbliche! Il decreto sui pagamenti della pubblica amministrazione, da voi tanto decantato, non considera adeguatamente gli enti in modo sano e virtuoso, che oggi in Italia si ritrovano nella paradossale situazione di essere esclusi da questi benefici; così, chi si comporta in modo efficiente, subisce più di altri i vostri tagli orizzontali! Siete riusciti, insomma, a far scomparire, ma solo per tre mesi, l'aumento dell'IVA. Avete sospeso l'IMU. State tergiversando sulla TARES. Gli italiani fiduciosi sperano dunque in una magia ben maggiore: che sparisca questo Governo! Per quanto riguarda le «misure straordinarie per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale», si può dire che il titolo del decreto è bello, ma solo il titolo. Secondo voi, misure che incentivino l'assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, in cambio di una decontribuzione pari a ben un terzo della retribuzione lorda, risolveranno davvero il problema ben più ampio di una disoccupazione che ha raggiunto ormai

è che quasi nulla si è trovato in questo provvedimento,

Costituzione sancisce che «L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro». È il primo articolo, non un articolo inserito nel corpo della nostra Carta costituzionale. No,

dalle politiche economiche l'economia. Oggi siete riusciti a rovesciare questa sequenza: oggi dall'economia (poi vedremo anche quale) vedremo anche quale) dipendono le politiche economiche; da queste, i diritti e i doveri del lavoro. Siete riusciti a far dipendere il lavoro dagli altri; il lavoro, da principale che era, è divenuto consequenziale. Quale economia, ci siamo detti prima? Se fosse basata quantomeno sull'attività economica - quella reale, quella dell'impresa con i suoi artigiani, imprenditori, lavoratori dipendenti, con le loro esperienze, macchinari, fatica, sudore sarebbe una naturale propensione al benessere dei suoi attori. Saremmo ancora nell'alveo delle tre funzioni sociali, su cui le comunità umane devono reggersi: funzione dell'attività economica, funzione politica e funzione culturale. Qui siamo succubi dell'economia finanziarizzata, quella che conta sull'incremento della ricchezza fine a se stessa, cinica, asettica, che si dirige verso un tornaconto individualista (che è molto diverso dall'utile individuale), che non guarda al benessere, ma alla speculazione. Il dominio dei mercati finanziari. L'ordine dei mercati finanziari. «Ce lo chiedono i mercati». Ce lo ricordiamo? «I mercati non capirebbero». «I mercati hanno bisogno». I cittadini hanno bisogno! I cittadini! Il popolo di lavoratori, imprenditori, artigiani, casalinghe, pensionati. E i nostri studenti. Sono loro che hanno bisogno. Noi, il Movimento 5 Stelle, siamo l'inizio, inarrestabile e irreversibile: mettetevi l'anima in pace. Siamo qui per ristabilire, riequilibrare e assicurare all'economia produttiva le risorse che la vostra economia, dominata dagli interessi finanziari, le sta sottraendo. Noi siamo la nuova liberazione, una nuova alleanza tra le tre funzioni sociali: economica, politica e culturale. Il provvedimento che ci accingiamo a votare avrà più pubblicità che risultati. È fuffa. È semplice melina. Vi serve esclusivamente per dare l'impressione ai cittadini che il Governo e la sua maggioranza (PD e PdL, sposi da sempre), stiano lavorando per il bene del Paese. Per il bene del Paese: una frase che vi esce dalle labbra più e più volte, come un mantra, che fate risuonare così tante volte che a un certo punto chi ascolta deve crederci. Per il bene del Paese. Non volete abbandonare il programma dei cacciabombardieri F-35, per il bene del Paese Non sfiduciate un Ministro diretto responsabile del Dicastero che ha consegnato una donna e una bambina di sei anni ad un Paese nel quale rischiano la loro incolumità, per il bene del Paese. Voi abusate della nostra intelligenza. Voi abusate molte e molte volte, e chissà quante altre ci aspettano. Il provvedimento che dovrebbe rivoluzionare il mondo degli occupati a tempo indeterminato offre risorse pressoché risibili: pressoché risibili: 500 milioni di euro per le Regioni del Mezzogiorno e 294 milioni di euro per le restanti Regioni. Il beneficio di cui trattasi si concretizza in una cifra massima di 650 euro al mese per massimo diciotto il calcolo è presto fatto: se tutto va bene, ossia se i legacci burocratico-normativi che sono presenti ancora nel provvedimento lo consentiranno, saranno appena 67.863 le unità lavoro che verranno occupate grazie a questo beneficio. Ma scendiamo nel particolare. Dati ISTAT:

iscritto a parlare la senatrice De Pin. Ne ha facoltà. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, le misure previste nel decreto-legge n. 76, che il Governo sottopone alle Camere per la sua conversione in legge, vanno a toccare molte materie. I provvedimenti che riguardano la promozione del lavoro giovanile, la riforma dei contratti precari, i tirocini e gli aiuti dati agli studenti, sia delle scuole superiori sia dell'università, pur andando nella buona direzione, hanno un difetto fondamentale: sono destinati a fallire perché non agiscono in profondità. Rappresentano purtroppo solo dei palliativi alla grave crisi economica e sociale che attanaglia il nostro Paese. A proposito di giovani e occupazione, questi sono alcuni dati diffusi dall'OCSE nell'ultimo Rapporto annuale sul lavoro nei 34 Paesi membri. Per quanto riguarda l'Italia,

nel nostro Paese è aumentata in modo preoccupante la quota di giovani *under* 25 che non lavorano e non vanno a scuola, la così detta generazione NEET, cresciuta di 5 punti percentuali arrivando fino al 21,4 per cento. Tra i Paesi OCSE, fanno peggio di noi solo la Grecia e la Turchia. Cifre preoccupanti, che ci mettono di fronte alle nostre responsabilità. Qualcosa dunque va fatto per cercare di risolvere questo drammatico problema. un Paese senza crescita dare lavoro ai giovani? Nel nostro Paese stanno aumentano vertiginosamente le ore di cassa integrazione e sono numerose le aziende costrette a chiudere e licenziare i loro dipendenti o a sottoimpiegarli in nero, come avviene sempre sempre più spesso anche in quello che una volta era l'operoso Nord-Est d'Italia. Il recente giudizio negativo da parte dell'agenzia di *rating* Standard & Poor's sui nostri titoli di Stato e il loro conseguente declassamento preannunciano un futuro a tinte fosche per la nostra economia. Se questo Governo, appoggiato da una maggioranza mai vista nella storia della Repubblica, non interverrà in maniera più coraggiosa, c'è il rischio che queste misure di promozione dell'occupazione non servano proprio a nulla. Infatti, aziende con fatturati in calo e un'imposizione fiscale eccessiva non possono permettersi di assumere giovani lavoratori, anche in presenza degli incentivi governativi. Nessuna di queste misure ha infatti come obiettivo quello di rilanciare lo sviluppo. Voglio ricordare che l'occupazione, e non solo quella giovanile, si rilancia solo con la crescita. Il rinvio dell'aumento dell'IVA ad ottobre e le indecisioni riguardo all'IMU giustificano le critiche più feroci rivolte al Governo di procrastinare le sue decisioni a tempi futuri. La mancata adozione di una necessaria e urgente riforma fiscale, che preveda una diminuzione delle imposte sulle attività produttive (IRAP) e sul lavoro (IRPEF), denota la totale assenza di coraggio dell'Esecutivo presieduto dal presidente Letta. L'anomala maggioranza che sostiene questo pavido Governo è infatti costantemente tenuta sotto scacco dai miserabili ricatti che provengono ora dall'una, ora dall'altra parte politica. Questo decreto non è pertanto all'altezza della grave emergenza che sta vivendo il nostro Paese. Invece di dare incentivi per l'assunzione di nuovi giovani lavoratori, lo Stato, come richiesto dalle imprese da molto tempo, dovrebbe diminuire il prelievo fiscale

Ora che questi crediti non sono più disponibili, a causa della difficile situazione del settore bancario, dobbiamo inevitabilmente adottare misure più coraggiose per sostenere la domanda. Senza reddito non c'è domanda e senza domanda non c'è produzione di beni e servizi. Dobbiamo invertire questo circolo vizioso garantendo ai lavoratori italiani una maggiore capacità di acquisto: un reddito più elevato comporterà una maggiore domanda e pertanto un aumento della produzione delle aziende. La crisi, prima finanziaria, poi economica ed infine sociale, iniziata nel 2008 non deve essere la giustificazione di tutti i nostri mali. Il declino dell'economia italiana viene da lontano ed è la conseguenza diretta di almeno un decennio

Signor Ministro, signor Presidente, colleghi senatori, esprimerò solo brevi considerazioni nell'ambito del tempo concesso, focalizzando l'attenzione sugli aspetti contenuti nel provvedimento oggi in esame

di tutta l'eurozona, con una percentuale di disoccupazione pari ad 11 punti, dato che cresce in Italia. Nel nostro Paese, i dati pubblicati di recente dall'ISTAT lanciano l'allarme in materia di lavoro: assistiamo con preoccupazione ad un'impennata del tasso di disoccupazione, che supera il 12 per cento, raggiungendo il livello più alto dal 1977 ad oggi. Si tratta di medie nazionali, che riassumono la condizione del Paese, ma tali cifre, in particolare, sono più gravi se vengono considerate regionalmente: al Nord il livello di disoccupazione è pari al 9,2 al Centro tocca l'11 per cento; nel Mezzogiorno sale al 20 per cento. Si tratta di una vera e propria crisi sociale che non consente alle famiglie di potersi costruire con certezza il proprio futuro. L'indice di disoccupazione giovanile, che si riferisce ai giovani tra i 15 e i 24 anni di età, si attesta al 40 per cento e scatta una fotografia ingiallita che evidenzia la mancanza di impiego delle nuove generazioni:

Come ricordato dal ministro del lavoro Enrico Giovannini, la carenza di occupazione delle fasce suddette costa ogni anno all'Europa 155 miliardi di euro, per via di un'assenza di utilizzo delle risorse umane. Nel dettaglio, in Italia si polverizzano 25 miliardi. Mi riferisco al fenomeno dei NEET, cioè a quei giovani che non ricevono istruzione e formazione. Parlando della crisi economica, anche Papa Francesco, giunto in Brasile ieri per celebrare la Giornata mondiale della gioventù, sottolineava che corriamo il rischio di avere un'intera generazione che non ha avuto lavoro e, in più, che dalla possibilità di guadagnarsi il pane deriva la dignità della persona. Ecco perché sviluppo e occupazione sono oggi più che mai le sfide da affrontare e i nodi da sciogliere per realizzare una società moderna in cui tutti, uomini e donne, e *in* *primis* i nostri giovani, possano avere le stesse *chance* che consentano loro di tracciare un percorso di affermazione delle proprie aspettative di lavoro. In relazione al provvedimento in esame nutro però delle perplessità sull'effettiva efficacia dello stesso e sulla capacità di offrire risposte adeguate in questi vortici di crisi globale. A tale riguardo, ritengo che il limite massimo, fissato a 29 anni di età, per usufruire degli incentivi previsti dall'articolo 1 sia troppo basso per consentire un *feedback* congruo e conveniente alle esigenze lavorative odierne. È risaputo infatti che la fascia di età tra i 18 e i 29 anni esprime una parte del tessuto occupazionale italiano e non risulta essere, tra l'altro, la più rappresentativa. Altra perplessità riguarda l'incentivo, pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per i nuovi contratti a tempo indeterminato, che rischia di non avere il giusto impatto sul mercato del lavoro, e questo perché le imprese oggi, come è noto a tutti, a causa della crisi economica sono nelle condizioni di licenziare i dipendenti in organico e non già di assumerne di nuovi. Terza perplessità: in merito all'imprenditoria giovanile l'Italia è in affanno sull'accesso al credito, troppo accentuato rispetto alle realtà europee ed internazionali. Per un giovane che ha un'idea imprenditoriale brillante... *(Richiami del Presidente).* Consegnerò il testo, perché non lo posso tagliare. *(Applausi

Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in questa situazione di grave crisi economica che tocca il nostro Paese e che coinvolge imprese, cittadini e lavoratori, ci viene chiesto un impegno straordinario Il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga è un grido di allarme lanciato dalle Regioni e riguarda tante situazioni individuali a cui dobbiamo far fronte. Dai primi dati, lo sblocco dei 550 milioni previsti nel decreto-legge n. 54 del 2013, che abbiamo convertito in legge lo scorso mercoledì, sebbene vada nella direzione auspicata, non basta. Ad esempio, nella mia Regione, la Toscana, sono stati assegnati 36 milioni di euro, che hanno consentito di coprire le necessità di 2.897 lavoratori. Rimangono però esclusi da copertura, secondo i dati della Regione, ancora 19.000 persone. Tutto ciò crea situazioni di tensione sul territorio, come è avvenuto con l'occupazione, seppure pacifica, del Comune di Scandicci da parte dei lavoratori dell'Elettrolux (ex ISI), preoccupati per una loro esclusione dalla CIG. Ma questa situazione non riguarda solo la Toscana. I dati del rapporto di giugno dell'osservatorio della CGIL parlano di oltre 530.000 lavoratori in cassa integrazione a zero ore nei primi sei mesi di quest' anno, e tutte le Regioni chiedono all'Esecutivo uno stanziamento ulteriore di 1,4 miliardi di euro per coprire almeno i fabbisogni dell'anno. Credo che si possa ad oggi valutare positivamente la sensibilità del Governo, che si è impegnato a finanziare gli ammortizzatori sociali e a garantire una efficace copertura integrale del fabbisogno dell'anno in corso accogliendo in Commissione, in sede di discussione di questo decreto, l'ordine del giorno a mia prima firma. Signor Presidente, colleghi, so bene che il finanziamento della cassa integrazione non è una misura risolutiva per la ripresa economica e il rilancio del Paese, ma sappiamo anche che a fianco dei provvedimenti per la crescita dobbiamo adottare provvedimenti incisivi per garantire la tenuta sociale, che altrimenti rischia di evolvere e passare dalla sfiducia alla protesta o, ancora peggio, alla rivolta. A questi drammi dobbiamo però rispondere prontamente sia con politiche di cura e di sostegno che con politiche industriali e di rilancio degli investimenti. Il primo investimento che facciamo con questo provvedimento è quello di credere nei giovani favorendo un loro veloce e qualificato inserimento nel mondo del lavoro e garantendo così alle imprese la possibilità di innovare e rendersi competitive. I provvedimenti per la tenuta sociale e per la crescita sono le due priorità la crescita sono le due priorità che dobbiamo portare avanti di pari passo per restituire fiducia e speranza, senza le quali difficilmente riusciremo a rilanciare il Paese e attrarre investimenti.

Presidente, sono Giuseppe, un cittadino, uno dei tanti che ha superato i trent'anni e - ahimè - ha perso il lavoro. Uno dei tanti che non ha voce a sufficienza per urlare la propria indignazione, la propria rabbia, la propria impotenza. Uno che ha la casa di proprietà, la prima casa, acquistata con il mutuo e che non riesce a pagare le spese condominiali, e allora...pignorano lo stipendio della moglie: 350 euro in meno ogni fine mese. Briciole per qualcuno che guadagna 14.000 euro, magari pagato solo per rappresentare se stesso. Uno dei tanti che ha seriamente pensato al suicidio. Uno dei tanti che però ama la vita e che si commuove guardando un tramonto o ascoltando del *blues*. Uno dei tanti perseguitati da Equitalia. Uno dei tanti che si vergogna di essere italiano. Uno dei tanti che votava a sinistra. Uno dei tanti che ora, in questo momento, ha bisogno di aiuti concreti, tangibili, facilmente misurabili. Uno dei tanti che ti chiede di raccontare che quando si perde la dignità, si perde anche un po' di libertà: libertà di movimento, di socializzazione. Uno dei tanti sfiniti di essere presi in giro. Uno dei tanti che mette 10 euro di benzina quando li ha». Ecco una *mail*, una delle tante. Signori, è un dovere dar voce a chi sta subendo tutto ciò. E non è un caso a sé, statene certi: lui, come tanti altri, è il risultato delle politiche fallimentari subite fino ad oggi. L'ascensore sociale non è solo fermo, ma è guasto, bloccato dal malaffare e dal malgoverno. Senza libertà materiale non c'è libertà politica né democrazia. Signori, non nascondetevi dietro un dito: l'Italia ha raggiunto 2.074 miliardi di debito pubblico, pari al 130,3 per cento del PIL, peggio di noi solo la Grecia. Cerchiamo di svuotare un oceano con un pentolino, ed è pure bucato! È la finanza a dettare tutte le regole! Se non sarà l'Italia a reagire, lo farà per lei il mercato con il suo linguaggio universale: ci sarà ci sarà un prossimo rialzo degli interessi richiesti, fino a rendere insostenibile il nostro debito. Ma come facciamo a dare speranze ai ragazzi? Abbiamo provato a sottolineare, nella discussione del disegno di legge n. 890, che le politiche giovanili non possono essere blindate fino ai 29 anni, ma non ci avete ascoltati. Volevamo innalzare la soglia almeno a 35 anni, ma ci avete detto di no. È avvilente vedere le persone che cercano lavoro con disperazione, e saremo curiosi si sapere quanti sono i figli dei politici che si presentano agli sportelli dei centri per l'impiego! Avete idea dell'opportunità di lavoro degli individui *over* 30? Quale futuro offrire agli *over* 30? La via della disperazione? La via dell'emigrazione? No, signori, questi cittadini hanno diritto di trovare queste risposte in Italia! Noi del Movimento 5 Stelle citiamo sempre la Costituzione; noi crediamo nella Costituzione, la reputiamo bella; «La bellezza salverà il mondo», e non è un'idiozia. non può essere capita e amata se non si possiede una Costituzione interiore e non può bastare se non la si ha dentro, se non la si sente come parte della nostra vita quotidiana, della nostra coscienza e del nostro spirito. L'anima viene prima di qualsiasi legislatore e di qualsiasi Costituzione. Alla fine non sono neanche tanto le regole che dettano le politiche, quanto l'egoismo o l'altruismo. Nel decreto-legge in esame abbiamo giocato alla farsa degli emendamenti, che hanno portato via tanta energia a tutti noi, e li avete sistematicamente accantonati nel balletto delle Commissioni con il ritornello velocissimo del:

se hanno dai 18 ai 29 anni, se sono disoccupati da almeno 6 mesi, se non hanno fatto studi superiori o universitari, ma solo scuole dell'obbligo o professionali. Sono requisiti che ci ricordano gli anni del dopoguerra: allora il lavoro veniva richiesto, oggi dobbiamo inventarcelo. Unica osservazione: negli anni passati c'era la strana abitudine che quando lavoravamo almeno ci pagavano. E ogni riferimento ai 18.500 lavoratori volontari di EXPO è puramente casuale. Signori, vorremmo ricordarvi che in Italia ogni due ore muoiono tre aziende; quelle che non sono fallite sono state comprate e smembrate da acquirenti esteri e multinazionali; quelle che restano stanno pensando di delocalizzare. Chi "produce ancora", lo fa nei Paesi dove gli esseri umani vengono sfruttati e schiavizzati e i loro territori inquinati e distrutti, poi si mette spudoratamente il marchio *made in Italy.* Sono pochi gli industriali che conservano umanità e senso dell'etica. Quando rinascerà un imprenditore come Adriano Olivetti, che concepiva la fabbrica come luogo di lavoro e di crescita culturale, fino al punto di affiancare agli operai e agli ingegneri figure come poeti e scrittori? Ecco, solo allora usciremo dal buio! Questi sono gli anni dell'avidità. È il caos. Bisogna chiedersi dove vogliamo andare, in quale direzione, con quali risorse e in quale situazione di socialità.

è lo spalancarsi, è lo spazio della separazione in cui non si tocca il fondo, in senso stretto è il vuoto. Il vuoto oggi impera; il vuoto è la distanza tra questa politica e Giuseppe, che chiede aiuti concreti, tangibili, facilmente misurabili, e che non ce la fa più!

Qualcuno potrà dire: ma sì, si aumentano gli acconti. Ma, signori stiamo parlando di acconti calcolati sul lavoro delle persone che non hanno il lavoro; stiamo parlando di una realtà in cui per riuscire a dare una soddisfazione politica alla propria maggioranza si chiede agli italiani di pagare tasse sul lavoro che non è stato ancora fatto e che neppure ci sarà. Cosa si creerà con questo? Un ulteriore buco!

ottenuto difficoltà nei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, che sono sempre più a disagio trovandosi con bilanci che verranno chiusi forse nel mese di settembre (non lo sappiamo ancora perché lo Stato non ha ancora chiarito quanto metterà a disposizione e se onorerà gli impegni assunti negli anni con i Comuni);

Questo non fa parte della scelta di un Governo che si è definito - come ha fatto all'inizio - di cambiamento e di coraggio. Allora, si abbia anche l'onesta di affermare - come si osserva in 5a Commissione permanente che per finanziare questi decreti si vanno a rimodulare provvedimenti e leggi vecchi di qualche mese o, nel caso migliore, di qualche anno. Questo non è possibile e va detto agli italiani.

questo è un Governo che sta subendo le pressioni della finanza, questo è un Governo che sta dicendo agli italiani di pagare le tasse perché il risanamento è all'orizzonte. Ma quale risanamento, se i conti pubblici sono sempre più una voragine? Dov'è il risanamento se il lavoro non parte? *(Applausi della senatrice Bisinella).* Diciamolo chiaro e tondo: il risanamento si fa a partire dall'occupazione, creando il lavoro, non andando a dire alle persone: verrete assunte perché lo dice il Governo. Le imprese non riescono ad assumere persone perché non hanno il lavoro, non perché ci sono

pagando anche più tasse, investendoli poi per abbassare il costo del lavoro. Diamo questi soldi a chi fa attività produttive: si creeranno nuovi posti di lavoro. Questo è il sistema dell'economia, questo è il sistema che garantisce a tutti una ripresa,

No, signori, noi siamo assenti perché lo abbiamo deciso, per protesta rispetto a tale atteggiamento. Noi non condividiamo questo modo di fare della maggioranza, e lo vogliamo dire a tutti i cittadini italiani.

ai giovani non si danno soluzioni a tempo indeterminato con questo provvedimento, si dà un piccolo sostegno, sperando che vi siano assunzioni, assunzione che non arriveranno, perché il lavoro non c'è. Inoltre, si parla di misure a sostegno del Mezzogiorno: chi non è d'accordo? Se parte il Mezzogiorno d'Italia, certamente

non aumenteremo le tasse. E perché allora nel decreto-legge c'è scritto: incremento dell'acconto IRPEF e dell'IRES? Questo significa far pagare più tasse alla gente! Con l'incremento dell'acconto sugli interessi maturati sui conti correnti e sui depositi

il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea e nessuno avrà il coraggio di far cadere il Governo. In questo modo però gli italiani andranno a fondo. Questo è un Paese che ha bisogno di scelte coraggiose, non ha bisogno di un Governo che porti l'asticella delle soluzioni un po' più in là perché non sa come intervenire. Non stiamo giocando al gioco delle tre tavolette con gli italiani. L'impressione, caro ministro Giovannini, è che stiate giocando a rubamazzetto con il portafoglio e il futuro degli italiani, e noi questo non lo accettiamo.

il provvedimento che vi apprestate a votare, in cui non c'è traccia di elementi quali innovazione, ricerca, rispetto per il lavoro e per chi lavora, non solo non porterà occupazione (io temo, anzi, l'esatto contrario), ma renderà di fatto il lavoro precario nel nostro Paese una pericolosa normalità. Altro che coesione sociale! Se c'è una cosa che conosco bene è il mondo del lavoro, quello vero. Ho lavorato 25 anni in fabbrica, di cui 16 in una catena di montaggio. Quella esperienza mi ha insegnato che i lavoratori vanno coinvolti, rispettati, non isolati e ridotti a passivi prestatori di mano d'opera, anche perché - voglio ricordarlo - sono quelli che realmente producono la ricchezza, e spesso sono i soli a tenere veramente al loro lavoro e alla loro fabbrica. Per questo mi permetto di dire a quelli che pensano che riducendo i diritti e la dignità dei luoghi di lavoro si può forse creare lavoro che si sbagliano di Solo chi non sa realmente cosa significa lavorare a certe condizioni può pensare infatti, da un lato, di chiedere la Commissione d'inchiesta sulla sicurezza sul lavoro e, dall'altro, di avallare il lavoro precario e senza diritti. Come si può pensare che le due cose siano compatibili? Ma veramente qualcuno può pensare che un lavoratore possa difendersi e denunciare eventuali mancanze su un tema tanto delicato, in un momento così drammatico in cui il lavoratore è consapevole che dal giorno dopo può essere mandato tranquillamente a casa Vi è tanto difficile immaginare uno scenario di questo genere? Con la scusa della crisi, e magari anche con modi gentili, il datore di lavoro può chiedere di lavorare dieci ore al giorno, invece di otto, e senza aumento di salario. Mi sembra di sentirli, le solite cose: «Sai, c'è la crisi», «posso assumere un altro che mi costa meno», e così via. Ma non sono cose che già succedono in Italia? O vogliamo far finta di non capire? Ecco perché noi di SEL pensiamo che questo tipo di lavoro non porterà nulla di buono. Oltretutto, la storia lo dimostra. Per favore, togliamo di mezzo l'ipocrisia. È ora di finirla con le strumentalizzazioni. Avete provato a mettere lavoratori e generazioni contro. Avete provato a dire che la lotta di classe non esisteva più o, comunque, che erano cose del passato. Ma poi avete fatto finta di non accorgervi che la lotta di classe esiste ancora, ma a farla sono i padroni nei confronti dei lavoratori, che, a loro volta, sono rimasti soli, isolati. Infine, avete provato a dire che imprenditori ed operai stanno dalla stessa parte, sulla stessa barca. È pur vero che tanti piccoli e medi imprenditori, che sono prima ancora dei lavoratori, hanno subìto e pagato questa crisi insieme ai lavoratori,

È altrettanto vero, però, che tantissimi imprenditori in Italia chiudono le fabbriche e vanno a delocalizzare solamente per pura convenienza. Non credo che i lavoratori abbiano questa possibilità. Non possono scegliere di andare altrove e se gli conviene; anzi, se gli va bene, potranno usufruire di 750 euro di cassa integrazione. Ora, sento anche dire che qualcuno addirittura la vuole togliere, come se fosse colpa dei lavoratori, degli operai. Solo per dire che, se proprio qualche volta i lavoratori e gli imprenditori si sono per caso trovati sulla stessa barca, è solamente perché gli operai servivano per remare, e non per altro. Concludo soffermandomi su uno dei tanti emendamenti presentati da SEL e puntualmente bocciato da questo Governo. Mi riferisco all'emendamento all'articolo 7 con il quale si chiedeva che i lavoratori potessero decidere tramite *referendum* della propria condizione. cosa più naturale di questo mondo per chi ama la democrazia, e per giunta si può realizzare a costo zero, ossia nelle ore previste dallo Statuto dei lavoratori,

a quale altra categoria di cittadini viene negata la possibilità di esprimersi sulle proprie condizioni come succede ai lavoratori? Gli operai sono cittadini italiani, quindi possono godere della tutela delle leggi e della nostra Costituzione, al pari di tutti gli altri? La politica, che da anni fa finta di nulla, può continuare ad ignorare queste verità? Se le regole che valgono in fabbrica fossero estese alla società intera, avrebbe senso la politica? Secondo voi esisterebbe ancora la democrazia in questo Paese a queste condizioni? Allora ditemi qual è la colpa degli operai, perché ancora non l'ho capita.

Signor Presidente, signori Ministri, signori colleghi, la situazione del mercato del lavoro italiano si è notevolmente aggravata a partire dalla seconda metà del 2011, dopo la relativa tenuta del numero degli occupati nella fase iniziale della crisi. Secondo un'indagine della Banca d'Italia, nel 2013 solo un quinto delle imprese industriali e dei servizi con almeno 20 addetti si attende un'espansione del numero dei propri occupati rispetto ai livelli medi del 2012 e la metà, invece, prevede una contrazione di questo stesso numero. A farne le spese maggiori sono i giovanissimi e i giovani adulti, i quali trovano difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro o a rimanerci, sia per la caduta della domanda complessiva sia per la diminuzione del *turnover* occupazionale. In un contesto simile era doveroso agire a favore dell'occupazione giovanile e sarebbe stato auspicabile poter discutere oggi di provvedimenti capaci di incidere a fondo sulle dinamiche di assunzione dei giovani disoccupati. Nonostante il lodevole sforzo del Ministro di intervenire su una molteplicità dì aspetti riguardanti l'occupazione e la formazione al lavoro, dobbiamo rilevare che gli incentivi economici predisposti, sia per modalità di erogazione che per ammontare complessivo stanziato, avranno effetti neutri o assolutamente poco significativi nei saldi occupazionali. Su una platea di potenziali beneficiari di quasi 3 milioni di persone, i vincoli di finanziamento consentono di incentivare l'assunzione al massimo di 50.000 giovani lavoratori l'anno. Sempre meglio che niente, si potrebbe dire. Se non fosse, però, che il vincolo imposto di assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato (aspetto apprezzabile in linea di principio), nel contesto economico che descrivevamo in precedenza, fa pensare che l'incentivo sarà sfruttato principalmente da quelle imprese che, per il proprio andamento economico anticiclico, avrebbero comunque assunto nuova manodopera, con o senza incentivi. Continuando in questa riflessione, l'incentivo previsto dal Governo potrebbe quindi avere il merito non tanto di aumentare l'occupazione giovanile, quanto invece di promuovere il contratto a tempo indeterminato quale forma contrattuale principale nelle nuove assunzioni dei giovani. Sarebbe anche in questo caso un intento assai condivisibile e lodevole, ma che viene decisamente contraddetto dalle disposizioni previste all'articolo 7 dello stesso decreto, dove si procede, di deroga in deroga, ad eliminare vincoli normativi relativi ai contratti di lavoro più flessibili, rendendo di fatto più facile l'utilizzo improprio di forme contrattuali di precariato al posto di forme occupazionali più tutelate. La riforma del lavoro del ministro Fornero, pur discutibile quanto vogliamo, possedeva una sua struttura logica: modificare l'articolo 18 per rendere meno diffidente il datore di lavoro nei confronti del contratto a tempo indeterminato e, al contempo, introdurre norme antielusione per ostacolare l'uso distorto dei contratti di precariato. E i dati del secondo semestre del 2012 mostrano proprio segnali di ricomposizione della domanda delle imprese verso posizioni *standard* di lavoro dipendente a scapito delle tipologie contrattuali atipiche, in linea con gli obiettivi della riforma. Questa riforma, così come strutturata dal ministro Fornero, fu già dalla prima lettura al Senato nella scorsa legislatura oggetto di modifiche da parte dei partiti che allora sostenevano il Governo Monti e che oggi sostengono il Governo Letta, guarda caso sempre nell'ottica però di indebolire le tutele previste per i lavoratori. Le misure previste dall'articolo 7, in perfetta continuità con le politiche neoliberiste del precedente del precedente Governo, non solo contrastano, snaturandolo ulteriormente, l'impianto della riforma attuata appena un anno fa, ma appaiono anche in contrasto con l'intento supposto dell'articolo 1 di questo stesso decreto. Le agevolazioni previste dal decreto per le assunzioni a tempo indeterminato, già insufficienti, come sottolineato, rischiano di perdere ulteriormente efficacia in un contesto normativo che torna a semplificare l'utilizzo di forme contrattuali atipiche. Puntare su contratti flessibili o comunque facilitarne l'utilizzo non è certo la soluzione per risolvere i problemi dei nostri giovani e tantomeno lo storico dualismo italiano interno al nostro mercato del lavoro tra contratti che garantisco stabilità e quelli che generano precarietà. I giovani non hanno bisogno solo di un impiego, hanno bisogno di un percorso professionale che garantisca l'attuazione dei loro progetti di vita e che permetta una contribuzione ai fini previdenziali cospicua e costante. Altrimenti i giovani disoccupati avranno come destino quello di diventare adulti precari e, in seguito, pensionati indigenti. E se anche dovessero, dopo anni di difficoltà e precariato, raggiungere un meritato successo professionale, certo non potranno aspettarsi, per effetto del metodo contributivo, di ricevere un vitalizio anche lontanamente paragonabile a quelle pensioni d'oro che la Corte costituzionale ritiene intoccabili, a tal punto da ritenere incostituzionale il prelievo di solidarietà sulle pensioni superiori ai 90.000 euro lordi. Da una parte abbiamo gli intoccabili con i loro diritti acquisiti e salvaguardati; da una parte abbiamo i *manager* privati e pubblici con compensi di centinaia di volte superiori a quelli dei loro colleghi impiegati: è una forbice in continua espansione. Dall'altra abbiamo gli esodati, i non salvaguardati, i giovani disoccupati, i nuovi poveri. Non vorremmo scoprire che l'ingiustizia sociale è diventato un diritto acquisito di questa nostra società e che nulla si possa fare per contrastarla. Siamo convinti e fiduciosi che non sia così. Per cambiare però questa tendenza, sarebbero urgenti e necessarie politiche redistributive più coraggiose, volte davvero a ridurre le disparità sociali presenti nella società. Politiche strutturali e non provvedimenti tampone e sperimentali come la *social card*. Tuttavia, nonostante le osservazioni fatte, riconosciamo che nel provvedimento in esame non mancano aspetti positivi. Invitiamo la maggioranza a valutare senza pregiudizi i nostri emendamenti, che in molti casi sono stati proposti con l'intento di migliorare quanto ritenuto già buono.

a modificare l'articolo 7, quello che peggiora quanto fatto dalla legge Fornero e che aumenta ulteriormente la flessibilità del mercato del lavoro. Pensiamo sarà sufficiente che vi convinciate (sempre voi del Partito Democratico) per una mezz'ora di essere un partito di centrosinistra. Si inizia con mezz'ora al giorno

un problema? È un problema per la nostra società? La sostenibilità del nostro sistema di protezione sociale è stata finora affidata ad una raccolta fondi basata sulla solidarietà fiscale, solidarietà tra i lavoratori, sulle imposte ai consumi. Poveri, esclusi, disoccupati, ammalati, bambini, non autosufficienti ricevono aiuti con soluzioni alimentate da queste modalità, in una logica, spesso meramente amministrativa, del raccogliere e del redistribuire. Ma i tassi di povertà persistenti e in aumento condannano l'Italia, che pure ha un invidiabile sistema di protezione sociale, tra i Paesi meno capaci di trasformare in valore sociale le risorse a disposizione. La Costituzione non limita i potenziali della responsabilità al solo raccogliere e al solo distribuire: ingiustizie e disuguaglianze vanno ben oltre la capacità redistributiva dei fondi a disposizione. Quindi, non si tratta di redistribuire o ridurre, ma di far fruttare il capitale a disposizione. le istituzioni, dopo aver raccolto le risorse con la solidarietà fiscale, devono evitare che siano consumate da aventi diritto senza doveri. bisogna, a nostro avviso, riconsiderare la capacità del rigenerare, ed è una sfida che può essere affrontata da tutti noi nelle condizioni difficili nelle quali ci troviamo. Vedete, per noi il lavoro è dignità,

anziane ancora autosufficienti, il servizio civile, le molteplici forme di lavoro del volontariato sociale. Dobbiamo quindi ripensare lo Stato sociale, piuttosto, come un servizio stabile e universalistico, rendendolo più leggero, ma allo stesso tempo salvaguardandolo, utilizzando comunque criteri selettivi a favore dei più deboli. L'obiettivo si può raggiungere se si riflette nell'ottica di utilizzare le politiche sociali per far ripartire la crescita, mentre diminuire le risorse sia sociali che sanitarie

con i loro servizi, raggiungono ben 6 milioni di cittadini. Ridurre pesantemente le politiche sociali e, più in generale, il *welfare* vuol dire rinunciare a posti di lavoro diffusi sul territorio e accessibili ad una vasta platea di giovani e di donne, fino ai disabili. In Italia, l'occupazione femminile è ferma al 46 per cento, venti punti in meno rispetto a quella maschile; è più bassa che in quasi tutti i Paesi europei, soprattutto nelle posizioni più elevate e per le donne con i figli: una su tre, infatti, è costretta a lasciare il lavoro alla nascita del primo figlio, per carenza di servizi. La disparità di retribuzione, a parità di istruzione e di esperienza, raggiunge anche il 30 Sappiamo che una donna su cinque non lavora, e al Sud il tasso di disoccupazione è davvero elevatissimo. Per questo abbiamo predisposto un emendamento che va ad incentivare l'assunzione delle donne. Non si può quindi ridurre il *welfare* e far gravare sulle famiglie, e dunque sulle donne, i tagli al tempo pieno nelle scuole, alla non autosufficienza, ai servizi alla persona, all'infanzia e alle famiglie. Si devono supportare maggiormente le famiglie; sì, le famiglie sono considerate come il maggior ammortizzatore sociale. Sul tema dei disabili e del lavoro ritengo importante l'ordine del giorno del PD, di cui sono prima firmataria, accolto in Commissione, per rivedere la posizione espressa dal Dipartimento della funzione pubblica in merito alla sospensione dell'obbligo di copertura della quota di riserva, vale a dire dell'entità di lavoratori disabili che i datori di lavoro soggetti ad obbligo devono avere alle dipendenze. È stabilito dalla legge n. 68 del 1999. Vi è la richiesta di rivedere il parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica e prevedere, considerando anche la gravità della situazione economica e sociale nel nostro Paese, misure mirate, specifiche ed urgenti volte a promuovere l'incremento dell'occupazione stabile delle categorie protette, anche per contrastare forme di marginalizzazione aggravate dall'attuale contesto di crisi economica. Al riguardo abbiamo

Le politiche degli ultimi decenni hanno tenuto poco conto delle realtà sociali in movimento, limitandosi a gestire gli strumenti giuridici ed economici già esistenti, senza spingere sulla leva dell'innovazione e dello sviluppo. Non si è investito sul rendimento. Non sono state cercate soluzioni più capaci di affrontare il rapporto tra bisogni e risorse. A forme più efficaci di aiuto e sviluppo umano e sociale, si sono preferiti sistemi assistenziali di tipo ordinario, senza una prospettiva futura. Al contrario, la richiesta di aiuto aumenta ogni giorno e non tenerne conto vuol dire non dare risposte, accettare che la sofferenza diventi disperazione, abbandono, conflitto, sfiducia, che generano assenza di prospettive con tutte le conseguenze del caso. È importante sottolineare in questo settore. Detto questo, il disegno di legge oggi all'esame dell'Aula rappresenta un primo importante passo per il Governo al fine della predisposizione di misure urgenti e semplificate in tema di lavoro, in particolare per ciò che concerne i giovani, e di coesione sociale, in linea anche con le politiche e le iniziative assunte a livello europeo e con la situazione economica e sociale che sta che sta affrontando il nostro Paese. È importante anche quanto previsto all'articolo 3, la cosiddetta Carta acquisti sperimentale, che integra la *social card* e rappresenta una misura importante contro la lotta alla povertà minorile, a partire dalle famiglie più marginali rispetto al mercato del lavoro.

Senatore Puglia, questa non è "fuffa", questo è un aiuto concreto. L'efficacia del programma si misura confrontando i risultati raggiunti dal gruppo dei soggetti beneficiari. dispone un'estensione, nei limiti di 100 milioni di euro per il 2014 e di 67 milioni per il 2015, a tutti gli altri Comuni delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna

per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche. Signor Signor Presidente, gentili colleghi, si discute per l'ennesima volta di nuove ed urgenti misure a sostegno dell'occupazione, soprattutto giovanile; un provvedimento non più rinviabile e imposto dalla crisi economica ed occupazionale che sta investendo il nostro Paese. Consentitemi però di fare alcune riflessioni ed evidenziare alcuni aspetti. Per l'ennesima volta è stato predisposto un provvedimento *omnibus*, finalizzato cioè a disciplinare con la solita approssimazione settori e materie assolutamente eterogenee, con il risultato di un testo normativo che, al pari di molti altri, detta norme che andranno a compromettere i delicati e complessi equilibri degli istituti giuridici vigenti. Appare essere un provvedimento istituzionale istituzionale obbligato, che rende più marcata la riforma Gelmini, e non un intervento a favore di quanti si trovino in difficoltà. Ad esempio, non possono non essere sottolineate le oggettive difficoltà del provvedimento nel disciplinare interventi a favore dei giovani frequentanti le scuole secondarie di secondo grado. All'interno del testo non sono state infatti previste norme di raccordo con l'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il successivo decreto legislativo 15

prescrive infatti, quanto segue: «I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale». L'obiettivo del decreto legislativo n. 77, quindi, è di far acquisire agli studenti, a partire dal quindicesimo anno d'età, con esperienze nel mondo del lavoro, soltanto alcune competenze professionali unitamente ad altre non necessariamente legate ad una professione o ad o ad una disciplina specifica, ma spendibili in diversi contesti e per finalità formative non paragonabili a quelle che si vogliono disciplinare con i commi 4, 7, 10 e 13 dell'articolo 2 dell'attuale testo in Aula. Si regolamenta la scuola e non il lavoro, si privilegia la formazione e non l'inserimento nel mondo del lavoro. Nel disegno di legge n. 890, invece, si vuole confondere il periodo di studio con gli interventi strutturati per l'apprendistato e con l'adeguamento delle abilità professionali per persone che nulla hanno a che fare con i banchi di scuola. Si dimentica forse che l'Italia soffre dal punto di vista occupazionale ormai da molti anni e discutere ancora in quest'Aula di una problematica, trasformata nel tempo in una vera e propria emergenza sociale, significa, signori, certificare il fallimento delle politiche di sostegno all'occupazione messe in atto nell'ultimo decennio, anzi nell'ultimo ventennio, dai Governi di qualsiasi colore politico posti al timone del Paese. Il tasso di disoccupazione si attesta al 12,2 per cento, in aumento di 0,4 punti percentuali rispetto a dicembre e di 2,1 punti negli ultimi dodici mesi. Sono stati spesi innumerevoli discorsi sulla necessaria conversione del nostro Paese ad un mercato del lavoro maggiormente flessibile, un'evoluzione presentata come propedeutica ai vertiginosi ed immediati aumenti dei posti di lavoro. La realtà che negli ultimi anni si è palesata, però, è del tutto opposta e può essere riassunta in un'unica parola: precarietà; precarietà del posto di lavoro che inevitabilmente si trasforma in precarietà della vita. Ma, paradossalmente, con la terribile crisi economica che stiamo vivendo, chi ha un'occupazione precaria può anche definirsi fortunato rispetto a chi non ha un lavoro o, come troppo spesso accade (anche in questi Palazzi), l'ha perduto. Tra i quindici-ventiquattrenni le persone in cerca di lavoro sono 655.000 e rappresentano il 10,9 In questa fascia d'età il tasso di disoccupazione, ovvero l'incidenza dei disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca, è pari al 38,7 per cento. Dati allarmanti che non possono più essere ignorati,

così come una diminuzione delle iscrizioni all'università. Questo sì che è davvero preoccupante per la cultura. Eppure non sono previsti neanche questa volta degli interventi di carattere strutturale, finalizzati a garantire una vera e maggiore occupazione, ma solo degli interventi Il presidente del Consiglio Letta, nei primi giorni del suo mandato, aveva fatto riferimento alla creazione di 200.000 posti di lavoro. Ora, ipotizzando l'utilizzo di tutti i fondi disponibili previsti dal provvedimento, si è ben lontani da quei numeri e anche dai 100.000 posti cui ha fatto riferimento il ministro Giovannini come risultato di queste misure. Gli stanziamenti previsti, infatti, sono 26 milioni per due anni più 28 milioni per il 2015 per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego ed altrettanti milioni per la realizzazione di progetti di infrastrutturazione sociale e valorizzazione dei beni pubblici nel Mezzogiorno, presentati dai giovani e dai soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate. Infine, solo 56 milioni di euro in tre anni per le borse di tirocinio formativo in favore di giovani dai diciotto a ventinove anni che non lavorino, non studino e non partecipino ad alcuna attività di formazione, ma residenti o domiciliati nelle regioni del Mezzogiorno. Il provvedimento in esame contiene inoltre misure con le quali si prevedono riduzioni del costo del lavoro, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, per l'assunzione di

L'esperienza passata ci dimostra però che gli incentivi alle assunzioni aventi carattere temporaneo sono del tutto inefficaci in quanto creano pochi posti di lavoro e ne beneficiano solo le imprese che farebbero comunque queste assunzioni. Sorge poi spontanea un'altra domanda: quale datore di lavoro decide di creare veri posti a tempo indeterminato, sulla base di un contributo pubblico che potrebbe non essere erogato, vista la limitata disponibilità delle risorse? Oltre Oltre queste criticità che ho evidenziato, non ho potuto fare a meno di notare nel testo la mancanza di riferimenti ad un territorio martoriato come quello dell'Abruzzo, con un altissimo tasso di disoccupazione, al punto che il relatore ha dovuto aggiungere, al termine dei lavori in Commissione, una chiarificazione, che non era presente nella versione originale, elencando espressamente le Regioni destinatarie degli incentivi. Con quest'ultimo emendamento avete dimostrato di saper andare oltre le inutili passerelle. Auspichiamo che la strada intrapresa continui ad essere percorsa.

ci accingiamo a esaminare un decreto-legge che, nelle intenzioni del Governo e di tutta la maggioranza, dovrebbe ridare ossigeno a un mercato del lavoro infartuato. Qualche beneficio effettivamente ne verrà per l'occupazione: le nuove norme in materia di contratto a termine favoriranno certamente una maggiore fluidità dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro; l'azzeramento del costo contributivo per il lavoro giovanile migliorerà i conti delle aziende che stanno assumendo lavoratori in questa fascia di età (anche se difficilmente incoraggerà altre aziende - su questo concordo con la senatrice Blundo - a fare altrettanto con la senatrice Blundo - a fare altrettanto nel prossimo futuro, dal momento che la provvista è destinata a esaurirsi troppo presto e chi tardi arriverà non potrà goderne). Ma credo che in questo emiciclo tutti concordino nel ritenere (anche se non tutti nel dire apertamente) che questi benefici sono e si confermeranno davvero di entità troppo ridotta rispetto alla gravità della crisi che il nostro mercato del lavoro sta attraversando. Le nostre imprese stanno operando in una congiuntura di estrema incertezza riguardo al futuro prossimo, non riguardo al medio o al lungo termine: incertezza riguardo a se e quando ci sarà l'inversione di tendenza, l'uscita dalla recessione; incertezza circa le tendenze in atto nelle economie di colossi mondiali come la Cina e l'India; preoccupazione persino sul futuro del sistema economico‑monetario continentale di cui facciamo parte. Chi assume una persona oggi è molto più incerto di quanto lo fosse dieci anni or sono sul punto se il lavoro da far fare a quella persona tra un anno o due ci sarà ancora oppure no. La legge Fornero, entrata in vigore proprio un anno fa, ha avuto il merito, niente affatto secondario, di stabilire sostanzialmente una «tariffa» per il licenziamento individuale dettato da motivi economici: da dodici a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione. Ma anche il costo minimo di dodici mensilità per lo scioglimento del rapporto, a uno o due anni dalla sua costituzione, comporta un aumento del 50 o del 100 per cento del costo retributivo complessivo. Si può ben comprendere che gli imprenditori siano molto riluttanti a correre questo rischio, anche quando hanno bisogno di aumentare gli organici. Così come si può ben comprendere che due anni fa la Banca centrale europea, impegnata nel salvataggio del nostro debito pubblico, ci abbia chiesto uno spostamento della protezione del lavoratore dalla sicurezza nel rapporto, con alto costo di separazione, alla sicurezza nel mercato del lavoro. L'alto costo di separazione nel rapporto di lavoro è proprio quello che Marco Biagi chiamava il «disincentivo normativo» alla costituzione di rapporti di lavoro regolari a tempo indeterminato; un disincentivo il cui effetto è ingigantito dall'incertezza mortale che caratterizza la congiuntura economica attuale nel nostro Paese. Ed è proprio qui che noi oggi dovremmo intervenire per facilitare le assunzioni, anche soltanto con un provvedimento di carattere congiunturale, sperimentale, di portata limitata al tempo necessario per uscire dal *tunnel* della crisi. Dovremmo poter dire agli imprenditori: «Finché non saremo fuori dalla recessione, assumete pure tutti i lavoratori che vi servono, senza preoccupazione per il prossimo futuro: per due o tre anni, se le cose andranno male vi sarà consentito di sciogliere questi rapporti senza rischi giudiziali e con un costo di separazione di modesta entità ma ben predeterminato». Questa sì che sarebbe una boccata di ossigeno tonificante per tutto il mercato del lavoro. E sarebbe una misura acosto zero che potremmo adottare senza le angustie in cui abbiamo dovuto costringere l'incentivo economico previsto dal decreto in esame per l'assunzione dei giovani. Offerto con tanta (e pur giustificata) austerità, difficilmente questo incentivo economico indurrà centinaia di migliaia di imprenditori a procedere alle assunzioni di cui avrebbero bisogno con un contratto a tempo indeterminato, se temono che la situazione possa cambiare cambiare in peggio nel giro di uno o due anni (e abbiamo visto come questo timore sia legittimo, giustificato). Un incentivo di questo genere avrebbe un impatto tonificante sul nostro mercato del lavoro enormemente più ampio e più forte di quanto possa avere un incentivo economico limitato nel tempo. Ancora Marco Biagi osservava come l'incentivo normativo possa essere molto più efficace dell'incentivo economico.

Non certo la preoccupazione di privare i giovani della prospettiva di un rapporto di lavoro più stabile: oggi, in una situazione in cui il Paese sta perdendo 30.000 posti di lavoro al mese (1.000 al giorno!) e in cui la disoccupazione giovanile è quasi al 40 a 99 giovani su 100 parrebbe di toccare il cielo con un dito se per un triennio si offrisse loro la possibilità di un rapporto a tempo indeterminato regolato in questo modo. Non sarebbero certo loro i controinteressati a una misura di questo genere. I sostenitori della immodificabilità, anche a titolo sperimentale, della vecchia protezione della stabilità del lavoro oppongono un solo argomento, uno solo, non ce ne sono altri: quello del «piano inclinato». Non si può toccare, neppure sperimentalmente, la protezione della stabilità del lavoro, perché si sa dove si incomincia, ma non si sa dove si va a finire. Questo è l'unico argomento contrario che nei giorni scorsi ci siamo sentiti ripetere, qui in Parlamento e fuori, dai colleghi e dai militanti del Partito Democratico e da sindacalisti di diversi orientamenti. da che mondo è mondo, l'argomento del piano inclinato, della *slippery* *slope*, è il cavallo di battaglia non dei progressisti, ma dei conservatori di ogni credo e di ogni osservanza. Da che mondo è mondo, invece, è proprio di chi lavora per il progresso, in tutti i campi, il metodo sperimentale: si prova, si vede che cosa accade, se i risultati sono insoddisfacenti si cambia strada, altrimenti si consolida e si generalizza ciò che si è sperimentato. Ma è con questo metodo pragmatico, con il metodo del *try* *and* *go*, non con le contrapposizioni ideologiche, che riusciremo a cambiare volto a questo nostro mercato del lavoro asfittico e ingessato. A dire il vero, all'inizio del dibattito in Commissione avevamo avuto l'impressione che qualche cosa si stesse smuovendo, su questo terreno, nel Partito Democratico. Ci aveva dato questa speranza un emendamento presentato dalla collega Ghedini, che prevedeva, in via sperimentale e congiunturale, una sostanziale liberalizzazione del contratto a termine nei primi trentasei mesi del rapporto tra l'impresa e il lavoratore. Era un'apertura strana, perché in quel modo, per non toccare una virgola della disciplina del contratto a tempo indeterminato, si sarebbe prodotto l'effetto di rendere assolutamente normale l'assunzione a termine. L'ho rilevato nel dibattito in Commissione, osservando che, in omaggio al divieto di toccare, sia pure marginalmente, la disciplina del licenziamento, il Partito Democratico appariva disposto addirittura a far sì che il contratto a tempo indeterminato sparisse del tutto per i primi tre anni del rapporto fra l'impresa e il lavoratore, sostituito in modo sistematico dal contratto a termine. Ma, ancorché fosse per questo aspetto paradossale, sarebbe stata comunque una misura utile nella situazione gravissima in cui ci troviamo. Invece anche questa timida apertura si è totalmente persa per strada. Il Ministro del lavoro ha rinviato l'intervento su questa materia a settembre, auspicando un avviso comune delle parti sociali. Scelta, questa, che sembra corrispondere all'appello del segretario della CISL Bonanni, affinché il compito di correggere le rigidità del nostro diritto del lavoro sia lasciato alle parti sociali. L'auspicio è che il sistema delle relazioni industriali sappia superare le difficoltà che gli hanno impedito in questi ultimi due anni di esercitare le proprie prerogative su questo terreno. Ma deve essere chiaro che, se anche a settembre dovesse registrarsi un nulla di fatto sul terreno dell'intesa tra le parti sociali, non potrà essere ulteriormente rinviata l'opera di semplificazione normativa e di rimozione dei disincentivi normativi all'assunzione a tempo indeterminato. Su questo punto chiediamo - anche con un ordine del giorno presentato all'articolo 1 del decreto-legge un impegno preciso del Governo. A questo proposito va detto che una grave emergenza nell'emergenza è costituita dalle centinaia di migliaia rapporti di collaborazione qualificata come autonoma, ma in realtà di lavoro dipendente, dei quali la legge Fornero richiede giustamente la migrazione nell'area del lavoro subordinato regolare. Il problema nasce dal fatto che la legge Fornero ha fatto il lavoro soltanto a metà, conferendo efficacia alle regole poste in questa materia dalla legge Biagi, ma non delineando, sull'altro versante, un rapporto di lavoro sufficientemente flessibile, sottratto alle bardature normative eccessive, per poter accogliere in modo universale tutto il grande mondo del lavoro dipendente. Oggi la migrazione dall'area della collaborazione autonoma a quella del lavoro subordinato determina un aumento di costo per l'impresa, parità di retribuzione oraria lorda, tra il 40 e il 50 per cento, oltre a tutta la maggior rigidità che caratterizza l'area del lavoro subordinato rispetto a quella del lavoro autonomo. Così stando le cose, è evidente che ci troviamo di fronte a un bivio: o torniamo indietro, alla palude del dualismo fra protetti e non protetti nel mercato del lavoro, abrogando o sospendendo le norme di contrasto all'abuso delle collaborazioni autonome, contenute nella legge Fornero; oppure di quella legge portiamo a compimento il progetto, mettendo a disposizione di lavoratori e imprese - almeno in via congiunturale, sperimentale un rapporto di lavoro subordinato che non comporti lo *shock* economico e normativo di cui ho parlato poco fa. tendono gli emendamenti sull'azzeramento dell'impatto del costo del lavoro sull'IRAP e sulla riduzione drastica del costo di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella sua fase iniziale, che abbiamo presentato in Commissione e che abbiamo dovuto ritirare di fronte alla determinazione contraria che ci è stata opposta. Completare l'opera avviata con la legge del luglio 2011, oppure tornare indietro: questa è l'alternativa di fronte alla quale ci troviamo, la scelta che dobbiamo compiere, se vogliamo risolvere l'emergenza di quelle centinaia di migliaia di collaborazioni false-autonome che rischiamo di perdere per strada al 90 Questa è la scelta che oggi, con questo decreto, noi non compiamo. Non la compiamo, perché siamo paralizzati dal tabù dell'intangibilità della disciplina del rapporto di lavoro regolare a tempo indeterminato. Peccato: è un'occasione persa. La speranza è che almeno il dibattito apertosi in questa occasione ci aiuti a non perdere anche la prossima occasione, che auspichiamo si presenti nel settembre prossimo. Un'ultima notazione. Questa legge nasce ancora sotto il segno della complicazione e della illeggibilità per la grande platea di coloro che sono chiamati ad applicarla. È tutta tutta scritta dagli addetti ai lavori in un linguaggio astruso, infarcito di riferimenti ad altre leggi, che solo dagli addetti stessi è comprensibile (perfettamente in linea, per questo aspetto, con i precedenti del collegato lavoro del 2010 e della legge Fornero del 2012). Questo non può non costituire un pregiudizio gravissimo per l'effettività della legge stessa. Ce lo dice l'Unione europea con il *Decalogue for smart regulation* del novembre 2009: una norma che per essere capita richiede il consulente non può avere la virtù di influire direttamente sulla cultura, sul comportamento di milioni, in questo caso di decine di milioni di persone. Anche l'estrema complicazione della nostra legislazione in materia di lavoro - e non soltanto il suo contenuto vetusto costituisce uno dei problemi maggiori per il funzionamento del nostro mercato del lavoro, per la sua trasparenza, per la sua apertura all'imprenditoria straniera, di cui tanto il nostro Paese avrebbe bisogno. Su questo, come su diversi altri capitoli politico-programmatici, chiediamo al Governo Letta nel prossimo futuro un colpo di reni. Gli chiediamo il coraggio di progettare un diritto del lavoro chiaro, incisivo e leggero al tempo stesso, capace di ridurre e non di aumentare i costi di transazione tra imprese e lavoratori; capace, nella sua semplicità, di essere veramente universale, come il nostro diritto del lavoro oggi non è, se è vero che esso si applica soltanto a metà dei lavoratori dipendenti nel nostro tessuto produttivo. un diritto del lavoro capace di parlare non soltanto a consulenti del lavoro e sindacalisti, ma direttamente a imprenditori e lavoratori, che hanno diritto di non sapere niente di diritto del lavoro e, ciononostante, diritto a capire che cosa la legge in materia di lavoro dice; un diritto del lavoro capace di parlare non soltanto agli *insider*, ma anche e soprattutto agli *outsider*, non soltanto alle vecchie generazioni, ma anche e soprattutto alle nuove.